Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 30 giugno. Oggi pomeriggio l'Assemblea esaminerà il disegno di legge sull'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. La prevista mozione sulla sicurezza da minaccia cibernetica è stata rinviata ad altra data che sarà stabilita da una prossima Conferenza dei Capigruppo. Pertanto, il sindacato ispettivo, già calendarizzato per domani pomeriggio, avrà luogo nella seduta antimeridiana di domani. La prossima settimana verrà discusso il disegno di legge di semplificazione, già approvato dalla Camera dei deputati e collegato alla manovra finanziaria, per il quale si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi. Seguirà l'esame di ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri e la discussione delle seguenti mozioni, ed altre connesse: Carlino, sulla mancata ratifica della Convenzione dell'Aja sui minori; Divina, sulla dipendenza dai videogiochi d'azzardo; Rutelli, sui flussi migratori dal Nord Africa; Filippi Marco, sul servizio di trasporto ferroviario. Nella seduta pomeridiana di giovedì 30 giugno saranno poste all'ordine del giorno interrogazioni a risposta immediata al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. alle ore 9, è convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale e di un componente del Consiglio superiore della magistratura. La chiama avrà inizio dagli onorevoli Senatori.

Perché abbiamo bisogno di un'Autorità garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza? E come nasce la proposta di istituire tale figura? L'esigenza di affermare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso un organismo indipendente e autonomo, nasce dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, che innova profondamente la cultura dei diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti. Il modo, infatti, di guardare all'infanzia e all'adolescenza condiziona il modo di essere delle culture politiche, alcune delle più rilevanti scelte delle politiche pubbliche e il rapporto tra vita privata e vita pubblica. Così come questo punto di vista influisce non poco su come le generazioni hanno coscienza di sé, della loro autonomia e dei loro reciproci legami e responsabilità, dell'insieme delle politiche di *welfare* e dei rapporti familiari. A loro volta l'insieme delle idee che riguardano l'infanzia e l'adolescenza non possono essere colte isolandole dal contesto sociale. Esse sono connesse ai fenomeni economici, demografici, politici; hanno una storia, non sono costanti. La politicità delle questioni che riguardano la vita e le esperienze delle bambine, dei bambini e degli adolescenti consiste in questo intreccio e costituisce la chiave di lettura del rapporto tra le famiglie, le comunità e lo Stato. L'innovazione più significativa avviene nel XX secolo. Il secolo trascorso è stato chiamato il «secolo del bambino». La Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata da un numero di Paesi mai raggiunto da nessuna Convenzione internazionale, compresa l'Italia, ne è stata la sintesi più avanzata. il bambino e l'adolescente sono considerati persone a un certo grado di sviluppo: titolari dell'universalità dei diritti propri di ogni essere umano e con particolari bisogni e interessi che implicano una specifica tutela. Il modo in cui si è coniugato e si coniuga il rapporto tra pienezza della titolarità dei diritti umani e tutela è proprio sia della sfera della politica, e quindi delle politiche pubbliche, che del rapporto adulti-bambini a partire dal rapporto genitori-figli. Le bambine, i bambini e gli adolescenti sono figli, ma il loro essere non si esaurisce in questo rapporto con i genitori. I loro rapporti fondamentali, da quelli affettivi, relazionali a quelli cognitivi, interni alle famiglie, rappresentano una dimensione assolutamente prioritaria, ma non sufficiente, a esprimere interamente la loro vita. Conseguentemente i diritti dell'infanzia, dentro e fuori la famiglia, devono essere intesi quali doveri che riguardano la sfera pubblica, concepita come l'insieme dei luoghi in cui si sviluppa il senso della comunità, il cui primo nucleo è quello della famiglia. In un saggio Carlo Alfredo Moro scrive: «Anche prima dell'approvazione della Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia del 1989 l'ordinamento giuridico, e il costume, avevano incominciato a prestare una certa attenzione ai diritti di personalità del soggetto in formazione; a riconoscere che egli non era solo un figlio di famiglia in proprietà dei genitori, ma un'autonoma persona (...). La Convenzione ONU di New York - bisogna riconoscerlo - ha fortemente sviluppato una nuova e più pregnante attenzione ai bisogni del soggetto in formazione, non solo perché ha espressamente evidenziato accanto ai diritti individuali anche quelli sociali del minore (...), ma anche perché ha previsto interventi positivi di promozione a tutela di ogni bambino, con problemi o non. E una pedagogia dello sviluppo umano che viene proposta dalla Convenzione e pertanto essa si rivolge, e impegna, non solo il politico o il legislatore o il giurista, ma ogni persona che comunque ha relazioni con chi, attraverso un difficile itinerario maturativo, ha bisogno - per non perdersi - di un forte aiuto e sostegno». Queste parole di Moro indicano in modo limpido e incisivo quale sia l'asse della Convenzione e costituiscono la premessa per un adeguato rapporto tra la Convenzione e le politiche concrete, le leggi per l'infanzia e l'adolescenza, a partire da quella sull'Autorità garante, figura prevista proprio nella Convenzione e che per il nostro Paese è quanto mai necessaria in quanto una moderna concezione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza stenta ad affermarsi. In Italia, infatti, che è agli ultimi posti nel mondo per crescita demografica, persiste una concezione in cui, secondo le ricerche più avanzate, gli attori deputati alla cura del minore sono i genitori o altri familiari stretti e lo Stato interviene solo laddove la famiglia non basta a sé, secondo un modello residuale che non risulta essere scalfito nonostante i sintomi di crisi. Questo è il problema che ci troviamo di fronte; questo modello residuale di *welfare* impedisce di leggere i cambiamenti intervenuti nella vita delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, nelle famiglie, nell'economia, nel mercato del lavoro. Occorre superare questo modello. La base di partenza è costituita dalla vita delle bambine, dei bambini e degli adolescenti - pensiamo solo al peso dei vecchi e nuovi media e dal suo rapporto con le modificazioni profonde che sono intervenute nella vita familiare, nel nuovo ruolo delle donne e nella nuova configurazione dell'economia *post*-fordista in epoca di globalizzazione, dove il ruolo dell'istruzione decide la competitività di un Paese e il futuro di ogni bambino. La riforma del titolo V della parte II della Costituzione può e deve essere occasione per una valorizzazione locale dei diritti universali, i quali dovrebbero costituire la chiave di lettura della nuova ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni. I diritti dell'infanzia sono il tipico esempio di vincoli e limiti dei poteri. Il nuovo assetto costituzionale in tal caso non può che indurre a delineare maggiormente non già il minimo dei diritti, bensì i livelli essenziali delle politiche pubbliche per i diritti fondamentali delle persone minori di età. I limiti dei rispettivi poteri tra Stato e autonomie locali devono essere ristabiliti a partire dai diritti di persone non adulte che hanno bisogno di determinate tutele per potersi sviluppare pienamente, senza incontrare ostacoli intollerabili. Le politiche pubbliche devono orientarsi in una duplice e convergente direzione: tendere a delimitare tutte le forme di discriminazione connesse alle diseguaglianze che attraversano i versanti istituzionali e sociali - accesso all'istruzione, servizi, e sostenere i percorsi della costruzione dell'autonomia dei bambini e degli adolescenti. Tanto la rimozione delle diseguaglianze quanto la realizzazione dell'autonomia comportano scelte politiche nei vari settori, dalle politiche dei bilanci alla valorizzazione di atteggiamenti culturali che siano di profondo riconoscimento di ogni bambino e bambina, di ogni ragazza e ragazzo. Perché il nuovo assetto non acuisca le differenze sociali tra i bambini e quelle tra i bambini del Nord e del Sud, è necessaria una interpretazione del titolo V che aiuti a indicare priorità precise, essenziali, nutrite da valori, e produttrici di programmi, puntuali e graduali, di realizzazione. Questa interpretazione è possibile attraverso una vera e propria Carta dei diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti che individui - a partire dai loro diritti soggettivi e sociali - i livelli essenziali delle politiche. Il dibattito intorno alla figura dell'Autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza si deve inserire dentro questi grandi mutamenti, a partire proprio da un radicale cambiamento del contesto in cui il bambino cresce e in cui può investire su sé stesso e assicurarsi un futuro. Dal bullismo all'anoressia e alla bulimia, dall'aumento delle droghe alle violenze subite e agite, dalla pedopornografia a forme di sfruttamento nel lavoro, niente può essere affrontato se non attraverso un grande investimento sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, tenendo in estrema considerazione, anche con uno sguardo nuovo, proprio l'adolescenza. Come si è detto, l'istituzione dell'Autorità garante deve essere concepita come uno strumento per dare piena e completa applicazione all'articolo 18 della citata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, che impegna gli Stati «alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo», nonché alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. Mentre molti Stati europei hanno dato seguito a tale indicazione, in Italia non esiste ancora un'Autorità garante a livello nazionale, anche se non mancano esempi di tale figura nell'ambito di alcuni ordinamenti regionali. Il primo Garante nazionale per l'infanzia della storia nasce in Svezia nel 1809, con il compito di difendere i diritti degli individui dall'abuso di potere da parte dello Stato. Successivamente altri Paesi del Nord Europa ne seguono l'esempio: la Finlandia nel 1919, la Danimarca nel 1955, la Norvegia nel 1962. Da allora la figura dell'Autorità garante è stata istituita in oltre 40 Paesi. In Occidente è stata istituita in circa 30 Stati e anche in America latina. In Italia, in attesa della nuova legge, è mancata un'Istituzione nazionale indipendente a garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e la sua mancanza è stata, anche in tempi recenti, rimarcata dal Comitato ONU sui diritti dell'infanzia nelle «Osservazioni conclusive» indirizzate al nostro Paese. Sono sempre di più le Regioni italiane che hanno approvato una legge istitutiva di un'Autorità garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, le Marche, il Lazio, la Calabria, l'Emilia-Romagna, la Campania, il Molise, la Puglia, la Liguria, la Provincia autonoma di Trento, la Lombardia, la Provincia autonoma di Bolzano, la Basilicata, l'Umbria, il Piemonte, la Toscana, la Sardegna, anche se ancora in molte di esse non sono ancora stati nominati i Garanti. Il disegno di legge, che giunge ora nell'Aula del Senato per la sua approvazione definitiva, dà finalmente attuazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo istituendo una Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Si tratta di un'iniziativa che discende da quella nuova cultura dell'infanzia e dell'adolescenza di cui ho parlato in premessa e che ha segnato una nuova e più attenta considerazione dei bisogni del soggetto in formazione. L'Autorità, che il disegno di legge propone di istituire, è caratterizzata da una posizione di indipendenza, da un forte rapporto con il territorio, dalla previsione di una consultazione attiva dei bambini e degli adolescenti, dalla partecipazione delle organizzazioni riconosciute dall'ONU e si ispira al principio di sussidiarietà, nel senso che rappresenta un ente facilitatore per l'affermazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Per una buona legge sull'Autorità garante erano necessarie tre condizioni: che il testo di legge fosse frutto in primo luogo del lavoro parlamentare, che il testo rispondesse ai criteri di indipendenza e di autonomia, con risorse finanziarie e umane adeguate, e che chiamasse a raccolta le migliori risorse associative, a partire proprio da quelle dei bambini e dei ragazzi, e quelle territoriali. La condizione migliore per la legge istitutiva dell'Autorità garante è che fosse il frutto di una vera convergenza. Il Governo Prodi aveva favorito il dialogo, permettendo, nonostante un testo proprio, alla Commissione parlamentare per l'infanzia, di cui allora ero Presidente, di elaborare un progetto condiviso. L'unica condizione posta era che la proposta venisse licenziata in tempi certi. Questo avevamo fatto e il testo era già stato inviato alla Commissione affari costituzionali di Camera e Senato. Il ricorso alle urne impedì poi l'approvazione della legge. Ma il metodo era quello giusto. E questo metodo produsse una linea condivisa in Parlamento e fuori. Si doveva ripartire da quei contenuti o perlomeno da quel metodo, o seguire maggiormente le indicazioni dell'Accademia dei Lincei. Questo percorso, dopo le significative incertezze iniziali, è stato poi ripreso dal ministro Carfagna con duttilità e attenzione. Oggi è un voto molto importante perché dice con chiarezza che l'Autorità garante dell'infanzia deve essere una Autorità garante vera e non può essere sottoposta ad altri poteri. L'Italia, come tanti altri Paesi, è preoccupata da vecchie e nuove forme di disagio dei bambini e degli adolescenti, ma rispetto agli altri Paesi lo dovrebbe essere di più per la povertà minorile, per nuove forme di esclusione, di abbandono scolastico. L'Italia, quindi, più di altri Paesi ha bisogno di un grande lavoro di un'Autorità di garanzia ben strutturata, in grado di tutelare e promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e stimolare tutte le amministrazioni e le istituzioni perché svolgano al meglio il loro lavoro. Ma occorrono strumenti e risorse adeguati e soprattutto saper mettere in moto dei processi al fine di stimolare le migliori energie del Paese. Questo deve fare l'Autorità garante e per questo deve essere indipendente da chiunque e richiamarci tutti a maggiori responsabilità verso i bambini e gli adolescenti. Per legiferare correttamente su un organo di garanzia come quello dei bambini, è necessaria la massima unità del Paese, al di là di ogni legittimo orientamento politico. Il lungo dibattito e la successiva approvazione in prima lettura del disegno di legge hanno consentito di individuare un punto di equilibrio per la costituzione di una figura centrale nel sistema di promozione dei diritti delle persone in età evolutiva, in sintonia con altre legislazioni europee. In particolare, i destinatari della tutela sono indicati come persone minori di età; l'Autorità garante detiene propri poteri autonomi di organizzazione e non è vincolata gerarchicamente e si configura come organo monocratico nominato d'intesa dai Presidenti delle Camere tra persone di notoria indipendenza, indiscussa moralità e specifiche e comprovate professionalità nel campo dei diritti dei minori. Devono poi essere sottolineati i rapporti dell'Autorità garante con l'iniziativa legislativa, in particolare attraverso il parere sul Piano di azione e di intervento per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, nonché le competenze relative alla collaborazione con organismi internazionali ed europei. L'Autorità garante, che presiede la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza composta dai garanti regionali o da figure analoghe, si pone come snodo essenziale tra i territori che presentano una variegata realtà di normative. Va ricordato, infine, che l'Autorità garante potrà segnalare alle procure della Repubblica competenti le situazioni che si configurino come disagio o abuso, competenza questa che ripropone il rilievo critico del confine con la giurisdizione. Il provvedimento si compone di 7 articoli, il cui contenuto richiamo in modo molto schematico. L'articolo 1 istituisce, al fine di assicurare l'attuazione e la tutela dei diritti delle persone di minore età, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica. L'articolo 2 disciplina le modalità di nomina dell'Autorità garante, organo monocratico scelto tra persone con requisiti specificamente previsti, con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. L'Autorità dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta. Vengono poi disciplinate le cause di incompatibilità e la determinazione dell'indennità di carica spettante all'Autorità. L'articolo 3 attribuisce all'Autorità garante una serie di funzioni di promozione, collaborazione, garanzia, nonché competenze consultive. Tra esse vanno ricordate la promozione dell'attuazione delle Convenzioni internazionali e della normativa europea e nazionale vigente; la collaborazione all'attività delle reti internazionali dei Garanti delle persone minori di a quella di organizzazioni e istituti di tutela dei loro diritti; la verifica della garanzia ai minori di pari opportunità nell'attuazione del diritto alla salute e nell'accesso all'istruzione; la formulazione di osservazioni e proposte circa l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi all'infanzia e all'adolescenza. Essa, inoltre, può esprimere pareri sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in tema di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; promuove le opportune sinergie con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e presenta alle Camere ogni anno - entro il 30 aprile - una relazione sull'attività svolta. Viene poi istituita, allo scopo di consentire la collaborazione con i garanti regionali, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'articolo 4 consente all'Autorità garante di richiedere informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori, alle amministrazioni e ai soggetti pubblici o a enti privati - nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza - nonché di accedere ed effettuare visite nelle strutture pubbliche e negli enti privati ove siano presenti minori. L'Autorità ha anche la facoltà di chiedere l'accesso ad archivi o banche dati, ai soggetti e per le finalità indicate. Tutti i procedimenti di competenza dell'Autorità si svolgono nel rispetto dei princìpi di cui alla legge n. L'articolo 5, in tema di organizzazione, istituisce l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, alle dipendenze dell'Autorità, con un numero massimo di 10 unità. L'articolo 6 consente ai singoli di rivolgersi all'Autorità garante per la segnalazione di violazioni o o situazioni di rischio di violazione, anche attraverso numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti. Spetta a una determinazione dell'Autorità garante medesima la definizione dei modi di presentazione delle segnalazioni e dei reclami che assicurino la semplicità delle forme di accesso. Infine, l'articolo 7 dispone sulla copertura finanziaria del provvedimento, quantificata in 1.500.000 euro a decorrere dal 2012 e in 750.000 euro per i sei mesi del 2011. Colleghe e colleghi, signor Presidente, signora Ministro, questo testo, come sappiamo, scioglie alcuni nodi importanti che hanno caratterizzato la storia della proposta per l'istituzione del Garante. Questi nodi erano relativi proprio alla natura e al ruolo del Garante stesso e riguardavano il rapporto con gli altri poteri dello Stato, con le organizzazioni della società civile e con le articolazioni territoriali. La delimitazione del ruolo si è avuta delineando l'azione dell'Autorità garante come azione sussidiaria rispetto agli altri poteri dello Stato e rispetto a un cambiamento delle funzioni delle autonomie locali dovuto alla modifica del titolo V. L'Autorità garante non è più vista quindi, come alcuni progetti di legge del passato, come parte dell'amministrazione o sottoposta al governo nazionale e locale, né caratterizzata da un'azione di denuncia aggressiva. L'Autorità garante svolge un ruolo sussidiario, nel senso che, a partire dal superiore interesse delle persone minori di età, agisce in modo attivo e responsabile per mettere in rete e coordinare le migliori energie del Paese. Chiama alla responsabilità perché essa stessa agisce con responsabilità. Il presente di oggi è già futuro. Il futuro degli uomini di domani è dato dalla cura dei bambini di oggi. Come dice un poeta: «Il bambino è il padre dell'uomo». L'investimento più lungimirante del Paese è dato dall'investimento sull'infanzia e l'adolescenza. Un Paese cresce se si investe su chi sarà protagonista del futuro del Paese. E un atto di generosità del Paese è quello di mettere al centro le persone minori di età. E' chiesto questo anche agli adulti, agli stessi genitori. C'è una frase di Gibran, ne «Il Profeta», che rende plasticamente il senso di questo, e con essa voglio chiudere Dice Gibran: «E una donna che al petto stringeva un bambino disse: Parlaci dei figli, ed egli disse: I vostri figli non sono vostri, sono figli e figlie della vita che solo di se stessa ha desiderio. Ne siete lo strumento, non l'origine. Anche stando con voi non vi appartengono. Potete dare loro il vostro amore, ma non le vostre idee. Hanno le loro idee. Date forse una casa ai loro corpi, non alle loro anime che stanno nella casa di domani che non entrerete neanche in sogno. Vi potete sforzare d'essere come loro. Ma non tentate mai di farli come voi».

Questo testo che istituisce l'Autorità garante per l'infanzia, come è stato già detto anche nella relazione e come abbiamo fatto fino alle ultime ore, è stato frutto di un lungo lavoro che va dalla precedente legislatura e che ha visto svolgere un ruolo fondamentale alla Commissione bicamerale per l'infanzia, ma - permettetemi di sottolinearlo - anche un ruolo significativo del PD nelle varie sedi istituzionali. È stato importante inoltre che ci sia stata la volontà comune di proseguire insieme anche dopo la battuta d'arresto che si è registrata in Aula alla Camera proprio su un testo, sul quale il Partito Democratico ed altre opposizioni avevano formulato osservazioni ed emendamenti proprio perché appunto vi erano in quel disegno di legge molti limiti da superare.

Il Partito Democratico ha messo con disponibilità a disposizione un patrimonio di proposte e di idee, ma anche il frutto di un lavoro di anni, di contatto con gli operatori del settore e soprattutto una visione ed un approccio sui diritti dei minori che ha visto sviluppare in Italia, a livello nazionale e locale, politiche sull'infanzia e sull'adolescenza

per la scarsa disponibilità economica di Comuni e Regioni. Oggi dunque più che mai nell'approvare questo testo sull'istituzione del Garante per l'infanzia (un testo che da anni

nonché una pratica e una cultura degli operatori del settore che in Italia ha dimostrato di essere molto avanti e molto qualificata sul piano delle competenze professionali.

relativo alla visione del minore, che ci fa uscire da un modello di protezione tutelare e che guarda al bambino, non più come soggetto incapace, solo da proteggere, non più come un *minus

Parte proprio da qui la premessa per l'istituzione del Garante e, come più volte abbiamo affermato, si è compiuto uno sforzo perché esso sia in sintonia con i principi della Carta di Parigi:

di protocolli d'intesa elaborati dagli ordini e dalle professioni, dalle amministrazioni locali, potrà esprimere pareri sul piano nazionale rispetto a provvedimenti sulla tutela dei diritti dell'infanzia

Tutto ciò, tutti questi diritti negati sono uno «scippo» al futuro, alla libertà, alla crescita delle persone.

una capacità di intervento, anche nei casi di violazione con segnalazione all'autorità giudiziaria. Finalmente diamo vita a uno strumento che potrà promuovere e vigilare sull'attivazione dei diritti universalmente riconosciuti: l'istruzione, la salute, la sopravvivenza, ma anche nuovi e moderni diritti, quale quello dell'identità legale, della *privacy*, della dignità e della libertà di espressione dei bambini e degli adolescenti. Vigileremo, con le nostre proposte, affinché un passo così importante nella direzione non sia contraddetto dalla sottovalutazione politica, programmatica e finanziaria che questo Governo ha adoperato nei confronti delle politiche per l'infanzia, per l'adolescenza e per le famiglie. Non è un caso che, a differenza di altri Paesi europei, l'Italia sia molto scoraggiata rispetto alla natalità. L'Italia invecchia e viene privata di un ricambio generazionale.

anche fortemente propositivi e collaborativi, affinché tutti insieme, al di là degli schieramenti, potessimo dare luce a questo provvedimento in tema di garanzie e dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

In questa occasione mi piace sottolineare e soprattutto ricordare che a partire dalla Dichiarazione di Ginevra del 1924 si è tentato di formalizzare

la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo) e in special modo più avanti, nel 1989, come ricordava la relatrice, con la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, che si assiste ad un vero e proprio cambiamento di rotta: si passa da una cultura che vedeva i bambini come oggetto del bisogno ad una che li vede come soggetti di diritti, al pari di qualsiasi altro essere umano. Tra l'altro, viene riconosciuto loro il diritto alla sopravvivenza, all'ascolto e a non essere discriminati e, soprattutto, viene affermato un principio base, quello del superiore interesse del bambino. Per la prima volta, inoltre, viene richiesto agli Stati non solo di riconoscere questi principi fondamentali, ma di farli propri. La stessa Convenzione costituisce infatti uno strumento giuridico vincolante per gli Stati che la ratificano, costringendoli ad uniformare le proprie norme a quelle da essa previste e anche ad attuare tutti i provvedimenti necessari ad assistere i genitori e le istituzioni nell'adempimento dei loro obblighi nei confronti dei minori.

È proprio in questi termini che deve essere anche letta la richiesta da parte del comitato di istituire a livello nazionale la figura del difensore civico per l'infanzia (garante, tutore, eccetera), richiesta peraltro ribadita dalla Convenzione europea sull'esercizio del diritti dei fanciulli del 1996 e dal documento conclusivo della sessione speciale delle Nazioni Unite del 2002.

insieme a lui i garanti regionali che sono altrettanto necessari perché assicurano la prossimità di questa figura istituzionale al territorio. In Italia, è stato detto, in attesa della legge, è mancata un'istituzione nazionale indipendente a garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e la sua mancanza è stata, anche in tempi recenti, rilevata dal Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nelle osservazioni conclusive indirizzate al nostro Paese. Come ricordava anche la relatrice, nel corso delle ultime due legislature sono state presentate numerose proposte di legge su questa materia e nella scorsa legislatura si è arrivati ad un testo condiviso che non ha visto l'approvazione per il ricorso

si istituisce l'Autorità garante che assolve alla funzione di promuovere una nuova cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, di vigilare sulla osservanza delle norme e di garantire il riconoscimento dei diritti dei minori. Il disegno di legge risponde all'esigenza di assicurare, in ambiti diversi da quello giurisdizionale, una tutela più ampia all'infanzia e all'adolescenza. L'intenzione è quindi anche quella di colmare il vuoto legislativo presente a livello nazionale con una legge che statuisca non solo l'istituzione di un'Autorità garante con poteri di carattere generale e di snodo relazionale tra gli organismi internazionali, nazionali e regionali, ma specifichi, altresì, una serie di indirizzi essenziali al ruolo dei garanti operanti in ambito regionale. L'istituzione dell'Autorità garante rappresenta un ulteriore tassello al mosaico delle politiche in favore dell'infanzia e dell'adolescenza ed uno stimolo necessario ad assicurare un «garante» dei minori radicato nella realtà territoriale in cui i problemi emergono, in grado di interloquire nella elaborazione delle politiche sociali,

a seguito del consolidarsi di una diversa cultura che vede i bambini e gli adolescenti non più come categoria a rischio, oggetto di tutela, bensì come cittadini portatori di bisogni specifici e soggetti di diritto. Il lungo dibattito, come diceva la relatrice, che ha fatto seguito all'approvazione della legge in prima lettura, ha consentito di sciogliere alcuni nodi e di individuare un punto di equilibrio per la costituzione di una figura centrale nel sistema di promozione dei diritti delle persone in età evolutiva in sintonia con le altre legislazioni europee. Rispetto al testo originario del Governo, la proposta ha ricevuto contributi rilevanti su punti qualificanti, tratti in particolare dal disegno di legge n. 811 presentato dal PD e di cui è prima firmataria la senatrice Anna Anna Serafini, tendenti a configurare l'Autorità, in sintonia con i parametri di Parigi, con i requisiti di indipendenza e autonomia. Un'attività dell'Autorità estremamente significativa, che merita di essere segnalata e meglio attenzionata, è quella della promozione della partecipazione di bambine, bambini e adolescenti alla vita delle comunità locali e del loro coinvolgimento nelle decisioni che li riguardano. Il tema della partecipazione alla vita amministrativa è già riconosciuto dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e rappresenta una nuova prospettiva culturale che aiuta a sviluppare una maggiore sensibilità all'ascolto ed alla comprensione dei bisogni e dei diritti dei bambini. Ad esempio, la progettazione partecipata di iniziative è la dimostrazione che è possibile accompagnare un esercizio significativo dei diritti e, al contempo, realizzare una comunicazione istituzionale tra la società adulta ed i minori. In conclusione, l'importanza e la delicatezza del tema ha richiesto una vasta e articolata consultazione che ha permesso di verificare «le priorità e le esigenze più avvertite nel campo della tutela dei minori», di «sentire la voce della società civile» nell'ottica di un più ampio riconoscimento della centralità del cittadino. Dietro questa proposta c'è stato un grandissimo lavoro anche da parte delle associazioni che si battono da sempre

del dibattito sulla tutela dei diritti individuali e collettivi dei minori. Appare, quindi, urgente l'istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, il cui ruolo è quello di far crescere soprattutto la consapevolezza, negli adulti e nei minori stessi, che i bambini sono soggetti titolari di diritti.

Paese ha ratificato, come tantissimi Paesi nel mondo, la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, ma la sua azione non è conseguente. Troppe sono le mancanze; avremmo bisogno di una svolta nella cultura dell'infanzia, nelle leggi e soprattutto negli investimenti. Penso, per esempio, al Piano nazionale per l'infanzia, privo di risorse e priorità, o al Piano nazionale per gli asili nido. La vita dei bambini, i loro bisogni, i loro diritti, il loro presente e il loro futuro devono diventare le priorità del Paese; le famiglie devono essere sostenute nella crescita dei propri figli. Per questo sono necessari un progetto lungimirante, un coordinamento delle azioni pubbliche e private e una valorizzazione delle competenze, perché

anche lungimirante l'investimento sul capitale umano e credo che l'investimento più efficace riguardi proprio i nostri bambini. Una politica che guarda lontano si sostanzia in nuovi investimenti per un *welfare* sostenibile, per servizi di qualità a sostegno

quello dell'infanzia è un tema che sta particolarmente a cuore a tutti. Proprio per questo, credo che il disegno di legge sarà discusso con estrema serenità, rispettandone il fine primo, ossia la piena attuazione e tutela dell'interesse dei minori, e rilanciando la cultura dei diritti dei bambini e degli adolescenti in tutti i suoi aspetti. Credo che quando riflettiamo sull'istituzione di una figura che faccia da autorità coordinatrice per l'infanzia e l'adolescenza e che sia in grado di tenere un filo conduttore tra le diverse esigenze che ci sono in questa materia non ci possano essere distinzioni di partito e connesse divisioni. Infatti, abbiamo lavorato tutti insieme in grande armonia. Questo provvedimento nasce grazie all'impegno del Ministro, nonché dal concorso di tutte le forze politiche che hanno dato il loro contributo; nasce con aspettative di grande valore. L'esigenza di assicurare all'infanzia una tutela più ampia di quella attuale e l'accresciuta consapevolezza negli adulti, e nei minori stessi, che i bambini sono soggetti titolari di diritto, hanno da tempo fatto emergere la necessità di procedere all'istituzione di un Garante nazionale per l'infanzia, figura già esistente in vari Paesi europei, come l'Austria, il Belgio, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, il Portogallo, la Spagna e la Svezia. si fa riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989, che prevede che gli Stati firmatari si adoperino per garantire i diritti del fanciullo anche attraverso la creazione di Istituzioni specifiche incaricate di vigilare sul loro benessere. In Italia, dopo la ratifica della Convenzione di New York, con la legge 23 dicembre 1997, n. 451, sono stati istituiti diversi organi per la tutela dei diritti dell'infanzia, a partire dalla Commissione parlamentare bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza, che ha compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali. La Commissione può richiedere informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività concernenti i diritti dei minori e riferisce alle Camere sui risultati della propria attività. Abbiamo poi l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, la cui Presidenza viene affidata congiuntamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche della famiglia. L'Osservatorio coordina amministrazioni centrali, Regioni, enti locali, associazioni, ordini professionali e organizzazioni non governative che si occupano della tutela dei diritti dei minori. è anche il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, che si occupa di raccolta e diffusione dei dati statistici, pubblicazioni scientifiche, predisposizione di schemi di rapporto, relazioni istituzionali; formula altresì proposte per l'elaborazione di progetti pilota e altri interventi. poi l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pedopornografia minorile, attualmente operante presso il Dipartimento per le pari opportunità, con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relative alle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni per la prevenzione e la repressione del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori. Diverse Regioni, com'è già stato ricordato in quest'Aula, hanno istituito con leggi apposite la figura del Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza o figure analoghe, poche però lo hanno effettivamente nominato, e speriamo che l'approvazione di questo disegno di legge possa accelerare i tempi per la nomina del Garante regionale in ogni Regione italiana. Manca quindi un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, che andrà a costituire una nuova struttura di coordinamento e permetterà finalmente di avere un quadro generale delle misure che si vanno ad attuare nei confronti dei minori. minori. Ovviamente non deve essere un sostegno in astratto nei confronti dell'infanzia, ma dovrà rappresentare se avere la forza e la capacità di raccordare e coordinare tutte le realtà regionali e - se vogliamo - tutti i garanti a livello regionale che verranno istituiti e quindi a coordinare e raccordare le varie organizzazioni che affrontano questo tema. Discutere del Garante per l'infanzia non è quindi cosa da poco, perciò dobbiamo essere grati al Ministro e a coloro che hanno calendarizzato finalmente questo provvedimento dopo venti anni d'attesa.

Signor Presidente, Ministro, colleghe e colleghi, faccia parte di quel movimento di "bambinisti" (scusate il neologismo che mutuo dal professor Scaparro che lo usa per se stesso per distinguersi dai "bambinologi", quelli che amano parlare dei bambini e fare poco per loro), per chi non faccia parte di questo complesso movimento (mi riferisco a quell'insieme di professionisti, educatori, associazioni e anche politici, soprattutto "politiche", come si vede anche dal dibattito odierno),

Al di là del fatto che il Sud del mondo ce l'abbiamo dietro l'angolo, e basta guardare (questo ci richiama all'analisi che faceva la relatrice, senatrice Serafini,

quando parlo dei problemi del Sud del mondo e dei pezzi del Sud del mondo che abbiamo in casa nostra, mi riferisco ovviamente ai ai problemi di bambini stranieri soli e quant'altro, usati per l'accattonaggio (le cose che sappiamo) e anche ad alcune questioni che riguardano gli italiani e che richiamava prima la collega Incostante. Questa sicuramente è una parte del ragionamento che non dobbiamo dimenticare. Al di là di questo fatto, si tratta di capire che con

ed incomincia un altro percorso, quello - come evidenziava la collega in precedenza - della costruzione concreta delle condizioni di esigibilità dei diritti dell'infanzia sanciti appunto dalla Convenzione ONU del 1989.

la funzione dell'Istituto degli innocenti per la raccolta, il monitoraggio, la diffusione delle buone prassi, che intanto incominciano a crescere nei Comuni con sperimentazioni, miglioramenti ed innovazioni

già detto e vi farò soltanto un accenno - è proprio il capovolgimento di un punto di vista: uscire da una cultura giuridica basata sul concetto di minore. Non è per un vezzo

il maggiore a cui è affidato il minore si riveli non in grado di occuparsene. Questo naturalmente è accaduto negli anni più recenti, perché c'è fior di letteratura che ci racconta come, in epoche nemmeno tanto lontane, non c'era neanche questa attenzione all'interno della famiglia, e ai minori succedevano cose anche certificate dalla legge. Peraltro, in Gran Bretagna è da pochi anni che sono state abolite le punizioni corporali come mezzo educativo nelle scuole. La

il minore è considerato per differenza rispetto all'adulto. Uno degli esempi più tipici - in uno degli ordini del giorno

di procedimento giudiziario, due tribunali diversi e due procedure diverse. Ciò per sottolineare come, nelle pieghe di una legislazione non messa a punto dal punto di vista della coerenza del diritto, ci siano ancora anomalie di questo genere. quindi di bambini e adolescenti come soggetti portatori di diritti propri, non derivati, da tutelare in quanto soggetti non autosufficienti e bisognosi di attività di cura, ma anche da promuovere. promuovere. La promozione dei diritti è forse l'attività più interessante affidata al Garante, nella sua autonomia: quindi, non un Garante interventista, che si sostituisce a a chi deve fare le politiche attive, ma un Garante che, assieme al monitoraggio, alla tutela, alla difesa, è anche promotore, stimolatore di iniziative sulla base di un'attenta lettura dei processi di trasformazione sociale, non solo in campo socio-sanitario-assistenziale o educativo, che sono i campi più ovvi e necessari, ma anche ad esempio su tutte le questioni delle politiche urbane che hanno a che vedere con le condizioni di vita generale del bambino. Possiamo fare un esempio: nella Convenzione delle Nazioni Unite si parla di diritto al gioco. Ebbene, ciò comporta da un lato un intervento sul fronte del lavoro minorile, perché i bambini devono andare a scuola e giocare,

del provvedimento al nostro esame, che è quella di favorire lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi i conflitti che coinvolgano persone di minore età.

*(PdL)*. Signor Presidente, colleghi senatori, signor Ministro, la storia dei diritti dei minori è una storia recente e nasce da un'evoluzione del concetto di «bambino», del modo in cui gli adulti lo vedono, del ruolo che di volta in volta gli assegnano nella società. Oggi sappiamo che un bambino è portatore di diritti, ma il posto occupato dai bambini nella nostra storia sociale è stato molto marginale, almeno fino a poco tempo fa, quando era un oggetto conteso tra i genitori, oppure un oggetto di sentenze senza contraddittorio. La prima svolta, da questo punto di vista, può collocarsi nel 1959, con la Dichiarazione dei diritti dell'infanzia che, in dieci principi, ha precisato gli obiettivi da perseguire per proteggere e aiutare i bambini. di un passo molto importante anche se, ancora, questa Dichiarazione considera il bambino come oggetto di cure e non come soggetto di diritto. Un salto fondamentale avviene nel 1989, con l'adozione da parte dell'Assemblea Generale dell'ONU della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia che, oltre ad essere un punto di arrivo, ha costituito anche un punto di partenza, o meglio di riferimento, per tutta una serie di iniziative legislative e operative, interne agli Stati o sovranazionali, a beneficio dell'infanzia. L'Italia ha ratificato la Convenzione sui diritti del fanciullo con la legge n. 176 del 1991. In questi anni sono state intraprese, successivamente, concrete misure di intervento per i bambini del nostro Paese. Ricordo, tra le altre, il Piano d'azione per l'infanzia e l'adolescenza del 1997, che nasce dal presupposto di promuovere i diritti di tutti i bambini, non solo di quelli in situazioni di disagio e di devianza, e l'istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia. La legge n. 149 del 2001 ha segnato una conquista in ambito processuale con la figura del «legale del minore» e garantendo l'ascolto del minore ultradodicenne in caso di giudizio. La legge n. 54 del 2006, poi, ha introdotto l'affidamento condiviso, che è divenuto la regola generale in caso di separazione dei genitori, col riconoscimento di un vero e proprio «diritto alla bi-genitorialità». Non mi sfugge né voglio nascondere che ci sono zone d'ombra in cui è necessario fare maggiore luce, affinare gli strumenti di intervento. Una di queste è l'estensione del lavoro nero minorile, in crescita soprattutto in alcune comunità straniere presenti sul territorio nazionale. Malgrado nel nostro Paese si possa realisticamente parlare di un indubbio successo dell'attuazione dell'obbligo scolastico, è stata ipotizzata la cifra di circa 200.000 minori, non suffragata da conferme ufficiali, bambini impiegati in lavori stagionali, per strada o presso parenti. Recenti inchieste riportano stime anche superiori, basate sul raffronto fra diversi indicatori, come l'abbandono scolastico, gli infortuni sul lavoro, la percentuale di bambini lavoratori all'interno delle comunità straniere, la crescente diffusione di forme miste scuola-lavoro. Mi auguro che il disegno di legge oggi in esame, che dà ulteriore attuazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo, sia anche la premessa per arrivare ad azzerare queste situazioni drammatiche. testo - come già detto dai colleghi che mi hanno preceduto - già approvato all'unanimità alla Camera ed attuativo della Convenzione sui diritti del fanciullo, discende proprio dalla nuova cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che si é affermata nel XX secolo, orientata dai principi messi a fondamento della Convenzione del 1989 quali: la non discriminazione tra bambini; il tenere sempre conto del superiore interesse del minore; la tutela del diritto alla vita e allo sviluppo dell'infanzia e, infine, ma non meno importante, l'ascolto delle opinioni del bambino in tutti i procedimenti che lo riguardano. Lungo è stato l'*iter* istruttorio in Commissione. Il confronto ha permesso la costruzione di un atto condiviso nell'interesse reale dell'infanzia. Ringrazio tutti i componenti della 1a Commissione per il lavoro per il lavoro svolto. Assieme all'impegno della relatrice Serafini, desidero ricordare quello profuso dalle colleghe del PdL, Allegrini, Rizzotti e Gallone, che, con l'ordine del giorno che verrà presentato e firmato all'unanimità, hanno collaborato a migliorare il disegno di legge rendendolo ancora più pregnante rispetto alle problematiche cui è riferito. Il provvedimento è stato trattato in Commissione con grande armonia e con esso si è veramente perseguito il bene comune.

rispondendo a questi nuovi indirizzi culturali che è chiamata a diffondere e difendere. La legge in discussione si caratterizza per essere ispirata al principio di sussidiarietà, nel senso che l'Autorità garante rappresenta un soggetto facilitatore per l'affermazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Proprio al fine di rendere la sussidiarietà concreta, ho proposto un emendamento affinché il Garante realizzi una propria autonoma programmazione pluriennale volta al raggiungimento di precisi obiettivi, nel contesto sociale del Paese, sulle linee di azione concreta che intende adottare,

anche altre necessarie per il miglioramento dell'atto medesimo, ritengo che essa possa trovare spazio nel previsto regolamento, che dovrà emanarsi entro tre mesi e che determinerà la struttura organizzativa e operativa dell'ufficio del Garante. In questo regolamento - mi sembra giusto suggerirlo - sarà opportuno indicare in maniera precisa le condizioni di incompatibilità dell'ufficio del Garante con altre funzioni ed incarichi, come quelli sindacali che mancano - per esempio - in questo disegno di legge,

più tempo di quello indispensabile, anche se l'atto - come ha detto la collega Adamo - è veramente importante ed è rilevante che tutti noi ci sentiamo coinvolti nella sua approvazione. Il regolamento acquista grande importanza alla luce della determinazione dei criteri di intervento del Garante nei processi civili, ma anche su quella che dovrà essere la modalità di costituzione e della composizione della Commissione consultiva presso l'Autorità. Occorrerà anche specificare in esso il rapporto sinergico, nel pieno rispetto della reciproca autonomia, con i Garanti regionali o delle Province autonome, sperando che non ci sia troppo burocrazia per ottenere risultati concreti e reali. Quest'ultimo è uno snodo delicato sul quale potrebbe giocarsi buona parte dell'incisività dell'azione di questa nuova Autorità, alla quale viene conferita dalla presente legge una serie importante di funzioni e compiti, concedendo anche diversi poteri di controllo e facoltà di intervento molto ampie. Tra questi sono certamente da sottolineare le funzioni di garante dell'attuazione dei principi costituzionali nell'ottica della tutela dell'infanzia e del soggetto in età evolutiva, nonché le competenze relative alla collaborazione con organismi internazionali e con gli organi centrali e periferici dello Stato. Viene tuttavia da chiedersi se, ad una mole così consistente di poteri, dei numerosi compiti, delle funzioni compiti, delle funzioni e - direi - dei doveri, si possa dare attuazione con una struttura che, al momento, è determinata da vincoli di organico e di bilancio non superabili, viste le finanze statali disponibili.

Il fatto è che nella società del benessere le problematiche dell'infanzia sembrano moltiplicarsi e non si può rispondere - come hanno cominciato a fare certe Regioni - solo con politiche di contrasto agli aspetti emergenti del disagio. Servono invece politiche per l'attuazione dei diritti, l'inserimento sociale, la cura specifica dei singoli casi, così come abbiamo previsto possa fare l'Autorità garante. prendendo a prestito le parole della relatrice, collega Serafini. Questa legge rappresenta veramente un punto di incontro felice tra diverse sensibilità ed orientamenti. Mi auguro però che possa essere felice soprattutto per i minori, perché più coinvolti nelle fragilità e nelle incoerenze di tanti adulti che troppo spesso dimenticano che un esempio è più utile di un rimprovero.

un tassello fondamentale per il riconoscimento dei diritti dei bambini intesi come persone e, quindi, autonomamente titolari dei propri diritti e non come minori oggetto di tutela. Molto bella è stata la citazione del poeta Kahlil Gibran con cui la senatrice Serafini ha concluso la sua relazione introduttiva, proprio per delineare l'identità del bambino autonoma rispetto a quella dei genitori e della propria famiglia. È importante che il disegno di legge che istituisce l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza sia di iniziativa parlamentare e sia nato da un percorso di condivisione che ha visto protagoniste tutte le forze politiche, partendo in particolare dalla Commissione bicamerale per l'infanzia.

quella di portare ad approvazione definitiva e di procedere all'attuazione dell'Autorità garante per l'infanzia e dell'adolescenza. È necessaria questa figura nel nostro Paese, più necessaria che mai, perché i diritti dell'infanzia, anche in Italia, anche nel 2011, sono negati, sono calpestati, sono non riconosciuti.

grandissimo nel nostro Paese: da un lato, troviamo le famiglie sempre più vicine, che accudiscono con sempre maggiore attenzione, che investono maggiormente sui propri figli, magari figli unici, che li accompagnano in un percorso sempre più carico di impegni e di aspettative;

a partire dal diritto ad una vita dignitosa (pensiamo, ad esempio, a tutti i minori non accompagnati che vengono nel nostro Paese), al diritto al gioco, al diritto alla salute, al diritto ad un'abitazione accogliente. Ecco, la povertà è legata all'infanzia. La povertà in Italia colpisce particolarmente le famiglie numerose, ovvero le famiglie monogenitoriali con dei figli; dobbiamo impegnarci perché questa povertà venga rimossa. E, ancora, il diritto all'istruzione, non ancora fruito adeguatamente nel nostro Paese: pensiamo che soltanto il 12 per cento dei bambini ha diritto all'accesso all'asilo nido; non tutti (purtroppo stanno aumentando) hanno diritto a frequentare la scuola dell'infanzia e, ancora, non hanno diritto ad una scuola sufficientemente accogliente e prolungata nel tempo. Basti pensare che il tempo pieno non si sta sviluppando e che il tempo prolungato quest'anno è drasticamente tagliato nelle nostre scuole.

che sono invisibili, in quanto non hanno un lavoro e non sono nella scuola: due milioni di ragazzi tra i 15 e i 24 anni che sono completamente spariti nel sistema sociale. Ecco, questi sono diritti negati. istituiamo la figura del Garante che è davvero molto importante; deve essere una figura indipendente, senza vincoli di subordinazione gerarchica, autonoma nella propria organizzazione; proprio per questo avremmo preferito che nella legge non fosse prevista solo la sua collocazione all'interno di una sede della Presidenza del Consiglio, ma che fossero fossero state legittimate altre sedi, proprio per marcare massimamente questa autonomia. Consideriamo però che la sede è un puro punto di appoggio organizzativo, non simboleggia alcun legame particolare con la Presidenza del Consiglio o con il Governo, proprio per valorizzare l'indipendenza e l'autonomia del Garante.

possa ascoltare le voci delle associazioni del volontariato, delle associazioni delle famiglie, dei rappresentanti dei soggetti che lavorano per la tutela dei diritti dei minori e i minori stessi. Sono bellissime le esperienze di consigli comunali dei bambini e degli adolescenti, nei quali i giovani direttamente presentano il punto di vista per il governo della città. Anche al Garante i bambini e adolescenti potranno presentare direttamente le proprie esigenze, i propri bisogni, ma anche le proprie straordinarie risorse, la propria creatività e la propria capacità di inventiva. Il Garante, quindi, deve essere un soggetto capace di grande ascolto, oltre ad essere anche lo snodo fondamentale di un sistema molto complesso, fatto di relazioni con i servizi delle aziende sanitarie, con i servizi sociali, con i magistrati e con coloro che tutelano i minori,

Paese. Credo che un ruolo fondamentale sia inoltre quello della promozione culturale, non solo per far emergere la violenza, lo sfruttamento e i pericoli che corrono i minori nella nostra società, ma anche per valorizzare la loro straordinaria capacità di costruire futuro. Per questa ragione penso che sia molto importante

perché il radicamento nelle comunità costituisce un elemento essenziale per il futuro dei bambini.

la figura del Garante per l'infanzia e l'adolescenza: una figura terza che deve essere autonoma e che sarà chiamata a promuovere ad ampio raggio la tutela dei diritti dei minori e a vigilare sull'applicazione in sinergia con tutti gli enti che operano in questo settore. Io mi auguro - questo voglio dirlo abbassando il tono di voce, però, spero con autorevolezza - che questa figura non cada nelle morse del burocratismo all'italiana. Altrimenti è come se avessimo perso un po' l'obiettivo per il quale stiamo lavorando e ci stiamo impegnando. Mi auguro quindi che questa figura di garanzia sia anche in grado di intercettare i bisogni i bisogni sia dei bambini e delle bambine, ma soprattutto della fase adolescenziale della vita che oggi si presenta come quella più problematica, quella verso la quale alcune volte il mondo degli adulti non è capace di cogliere i segnali che il mondo adolescenziale ci offre, al punto che essi diventano delle vere e proprie patologie.

Il Paese ha bisogno di investire sull'infanzia e sull'adolescenza perché è un Paese che invecchia. I dati che ci ha fornito l'ISTAT sull'invecchiamento della nostra popolazione sono eloquenti, ma anche molto, molto preoccupanti. Dobbiamo quindi avere - speriamo che ognuno di noi la abbia - la consapevolezza che si sta compiendo un passo importante perché la vera garanzia di tutela dei diritti dei minori, il vero riconoscimento delle pari opportunità di fanciulli ed adolescenti parte necessariamente da una politica di sostegno effettivo alla famiglia.

di mettere insieme le politiche per l'infanzia e l'adolescenza e le politiche per la famiglia, affinché ogni bambino abbia la possibilità, dopo la nascita, di continuare la sua crescita, il suo sviluppo ed anche l'avventura della sua vita proprio all'interno della famiglia. Come si può infatti parlare di diritti dell'infanzia se in Italia le famiglie vivono in una situazione di affaticamento? Alcune volte questo affaticamento supera la soglia dell'umana tollerabilità. Le famiglie si sentono abbandonate dalle istituzioni, soprattutto se i nostri giovani troppo volte vengono anche derisi. In fondo, i dati che l'ISTAT ci presenta dimostrano che nel 2010 la natalità è calata e ci sono state 12.200 nascite in meno rispetto al 2009. Nell'ultimo rapporto ISTAT, presentato il mese scorso, questo istituto di ricerca ha anche fotografato una realtà terribile. Un quarto degli italiani circa vive sulla soglia di povertà: le nostre famiglie, quindi, una parte consistente di esse. Questo è il tassello mancante. Io credo, quindi, che accanto alla figura del Garante, sia fondamentale dare attuazione ad una politica efficace per le famiglie, così da garantire loro non solo il minimo indispensabile, ma anche la possibilità di far crescere, di educare e di accompagnare i figli nelle scelte fondamentali della vita. L'approvazione di questo disegno di legge, quindi, deve essere accompagnata da questa consapevolezza unanime e condivisa: che il nostro lavoro non deve fermarsi qui, che questo è un primo passo al quale dovrà affiancarsi, nel minor tempo possibile, una politica fiscale a sostegno delle famiglie e, quindi, un reale sostegno anche per i bambini. Il Presidente del Consiglio, proprio ieri qui in Aula, ha ha detto che non vorrà far pagare alle generazioni future le difficoltà del presente. Speriamo, quindi, che ci siano delle politiche conseguenti in questo senso. Giuseppe Mazzini definiva la famiglia come la patria del cuore, noi oggi dobbiamo tutelarla e garantirla appieno. Voglio chiudere con due affermazioni. Una la mutuo da un padre della nostra Repubblica, Alcide De Gasperi, quando, in un suo discorso a Milano nel 1949, diceva che «politica vuol dire realizzare». Noi oggi stiamo mettendo un tassello nella realizzazione, ma sappiamo che che è solo un tassello di un *puzzle* più ampio. Se, invece di parlare noi adulti, avessimo fatto parlare i bambini, loro forse avrebbero usato un linguaggio diverso dal nostro. Avrebbero usato delle parole, però ci avrebbero stupito. Speriamo che, anche attraverso questa scelta, i nostri figli, di oggi e di domani, possano continuare e, ancor meglio, stupirci.

siamo faticosamente arrivati, con un po' di ritardo, e pare che la fatica non sia finita,

Presidente, desidero solo sottolineare all'Aula, e naturalmente alla Presidenza del Senato, la necessità che venga garantita dalla Presidenza stessa la continuità della seduta.

Signor Presidente, non mi faccia interloquire su questo piano, perché la Presidenza del Senato ha una composizione sufficiente a garantire la continuità

di sottolineare l'opportunità che la Presidenza del Senato organizzi i lavori in modo che la seduta possa svolgersi in modo continuativo, senza interruzioni.

cortesia istituzionale: qui si tratta soltanto di garantire i lavori dell'Aula. Questa mattina abbiamo anche sospeso i lavori in attesa che arrivasse il Ministro, che ringrazio per essere qui presente, e nessuno ha sollevato alcuna obiezione. Oggi ci troviamo nella condizione

Collega, i rapporti di cortesia istituzionale, che ci sono sempre tra la Presidenza e i Gruppi, sono notori: è accaduto tante volte che i Gruppi, per una riunione di direzione... GIAMBRONE *(IdV)*.

si possa e si debba convenire per il buon andamento dei lavori su un rinvio o su un aggiornamento. La notazione politica che le sottopongo riguarda però il complesso dell'attività del Senato. Penso non sia mai accaduto nella storia del Senato che di mercoledì pomeriggio

l'argomento che mi ero permesso di sollevare non riguarda il fatto che le si debba, sia a lei che ad un altro Vice Presidente che si trovi nella stessa condizione particolare, il gesto di cortesia e disponibilità

giornate nelle quali non si lavora nell'Assemblea, perché non c'è attività legislativa, non c'è attività di indirizzo, non c'è attività nella quale il Senato deliberi. Dunque, il fatto che vorrei sottolineare non è il dissenso su ciò che lei ha detto, cui affido invece consenso:

il Senato lavora sempre meno e legifera sempre meno. Questa è la fotografia che emerge oggi, e tanto credo fosse necessario dire. l'Aula lavora secondo il calendario del lavori che ho letto, proprio all'inizio della seduta, per la prossima settimana. Comunque, è un problema che non appartiene alla mia decisione in questo momento. Io seguo l'ordine del giorno che è stato concordato tra i Capigruppo o all'unanimità o a maggioranza.

Questo impegno l'avevamo formalmente preso in svariate situazioni, e me lo ricordo perché ho partecipato personalmente alla speciale sessione ONU sull'infanzia del 2002

con varie modalità questa figura: alla Svezia, che è stato il primo, se ne sono aggiunti molti altri. Ricordo poi il lavoro che ha portato a questo testo di legge, che parte da molto lontano, perché

dai colleghi e dalle colleghe. Credo sia importante rimarcare come venga messo al centro del provvedimento di legge il fatto

dal testo, del Garante per l'infanzia? Avrà una funzione di promozione culturale, quindi sarà una leva per produrre un cambiamento culturale negli adulti che hanno responsabilità verso i bambini; una funzione molto importante di ascolto dei minori e dei loro rappresentanti che servirà per comporre i conflitti, ma anche per monitorare, in linea generale, le quali i minori si trovano spesso a combattere. Parlo specialmente di quei minori che vengono allontanati dalla famiglia e accolti presso strutture d'affidamento, che sono particolarmente sensibili. avere una funzione di ricerca per incrementare le conoscenze e trovare il sistema di uno scambio di buone prassi, così da fare un lavoro di rete anche con tutte le organizzazioni che si occupano di minori: la Commissione parlamentare, l'Osservatorio nazionale, il Centro di documentazione, l'Osservatorio per la pedofilia, il Comitato per i minori stranieri, il Comitato media e minori, il Comitato adozioni internazionali e l'Osservatorio sulla famiglia. Li ho citati tutti, perché, in effetti, un po' c'è - purtroppo - il dubbio che ci sia qualche difficoltà nello svolgimento di una funzione di rete che non sovrapponga competenze. Vedremo nella pratica se si riuscirà a far sì che non vi sia un'effettiva sovrapposizione di competenze, ma piuttosto una collaborazione per arrivare alla alla finalità che è, appunto, quella della tutela del minore. È già stato citato un problema che penso il Garante contribuirà a risolvere: mi riferisco a quello della formazione. Voglio fare una notazione sul fatto che ritengo molto importante l'esperienza dei Garanti regionali. Le prime tre Regioni che hanno istituito il Garante sono le Marche, Marche, il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia (poi se ne sono aggiunte delle altre). È importante l'esperienza che è stata maturata nelle Regioni, anche perché sono poi sostanzialmente le Regioni che fanno il lavoro di programmazione di tutti gli interventi sul sociale. Quindi, bisogna assolutamente chiarire che i Garanti regionali non sono in una posizione di inferiorità o di dipendenza

possa influenzare positivamente anche tutta la discussione sulla riforma del diritto minorile. Sapete che si è posta anche nella XIV legislatura, e si pone ancora, un'importante questione sulla necessità di una riforma dei tribunali dei minori: se ne è discusso a fondo. Credo che il Garante per l'infanzia e l'adolescenza possa rappresentare una possibilità affinché non tutto quello che riguarda i minori debba essere giuridicamente risolto in un'aula di tribunale. Attraverso il lavoro che fanno anche i Garanti regionali si potrà dar luogo a a quel tipo di giustizia mite, che non è per forza la giustizia amministrata nelle aule dei tribunali e basta. Questo credo che sarà un fatto importante. So che sono stati presentati emendamenti (molti sono stati anche ritirati) e ordini del giorno. La speranza - lo ripeto - è che questo provvedimento porti all'istituzione di un'Autorità che sia competente, indipendente, capace

che, nella sostanza, a poco servono e nulla fanno del lavoro che spetterebbe loro. Mi auguro che nel caso del Garante per l'infanzia e l'adolescenza non sia così. Termino l'intervento con questo auspicio. Ripeto: ho qualche dubbio, ma saranno la pratica e l'istituzione che

a parte il fatto che non mi viene in mente nessuna delle autorità che non starebbe svolgendo il proprio ruolo nel migliore dei modi, occorrerebbe magari fare il ragionamento inverso: noi abbiamo creato, seguendo il modello anglosassone, le *Authority*, non abbiamo un modello anglosassone legislativo di riferimento, il che secondo me complica la vita alle *Authority* e anche ai cittadini che non possono godere in pari misura degli stessi diritti civili, politici, economici, sociali, culturali, o comunque dei diritti umani. Sicuramente, tra questi ci sono i fanciulli, che in questi ultimi mesi sono stati al centro di molti provvedimenti che abbiamo adottato, ma purtroppo - lo ricordava nel suo intervento anche la senatrice Incostante - non sempre la qualità delle politiche (in alcuni casi anche dei provvedimenti) ha dato l'esempio - visto che dell'esempio ci è stato detto occorre essere Non è sicuramente il tempo di fare delle polemiche. Nel dibattito alla Camera e anche in Commissione qui al Senato alcune di tali questioni sono state sollevate, però credo che molti degli aspetti che hanno a che fare con i diritti del fanciullo debbano continuare ad essere tenuti sotto grande considerazione ed attenzione. E molto probabilmente, proprio perché si è adottata la decisione

prendere in considerazione quel che non va e applicare magari le buone prassi straniere e anche alcuni ulteriori miglioramenti delle istituzioni che andiamo a creare quest'oggi. Con la senatrice Poretti avevamo presentato il disegno di legge n. 1855 che era un po' più aggressivo riguardo alle funzioni che il Garante avrebbe dovuto svolgere. Abbiamo cercato, allo stesso tempo, con quattro ordini del giorno, di affrontare alcuni degli aspetti che

che, ahinoi, ancora una volta occorre rimettere sotto un cappello unico, riorganizzare nel migliore dei modi possibili, perché appunto i tribunali devono trattare i cittadini italiani - e non solo italiani nello stesso modo. Vi sono molte proposte, tra le quali anche quella dell'ex ministro Castelli, che andavano in questa direzione e spero che i colleghi della Lega vogliano recuperarla per rimetterla all'ordine del giorno Un altro dei nostri ordini del giorno prendeva in considerazione la modalità di revoca dell'adottabilità: anche questo è uno dei problemi molto gravi, che secondo noi resta. E ci sono delle proposte di legge che potremmo utilmente recuperare anche dalle scorse legislature, dalle scorse legislature, come - in particolar modo nella XIV legislatura quella dell'onorevole Biscardini, che con la senatrice Poretti domani ripresenteremo - e ve n'è una relativamente alle sentenze di condanna della Corte europea, che producono delle enormi sanzioni economiche per l'Italia sempre nei casi di adozione, ma non consentono la revoca dei provvedimenti di adottabilità. Il problema della risposta dell'Italia dal punto di vista normativo oltre che politico nei confronti delle sentenze della Corte di Strasburgo resta tutto, indipendentemente dalle dichiarazioni del Governo. Abbiamo la fortuna di avere però qualcuno nel Dicastero deputato a tali questioni, la ministra Carfagna che è con noi e che ha voluto seguire tutto il procedimento fin dall'inizio, che è molto sensibile alla questione. Occorre però che alcune posizioni relativamente alla giurisdizione internazionale siano condivise con altri Dicasteri, che non sempre sono inclini a prendere in considerazione ciò che ci viene detto da Strasburgo.

per cercare di evitare che queste persone vengano considerate come dei tossicodipendenti "da strada" e quindi per non escluderle nei processi di affidamento dei minori a disposizione, o magari per recuperare il ruolo dei nonni - qualora vi siano - come persone alle quali poter affidare questi soggetti e quindi aiutare sia i bambini a rimanere con i genitori, sia i genitori ad intraprendere nel migliore dei modi possibili un percorso di fuoriuscita dalla dipendenza dalle sostanze stupefacenti. Nei mesi scorsi, sempre focalizzandoci sui diritti dei bambini, abbiamo adottato una legge, che purtroppo entrerà in vigore nel 2014, relativamente alle detenute madri, per andare incontro alle esigenze dei bambini. Speriamo, nelle prossime ore, di portare a termine la ratifica della Convenzione di Lanzarote, che ancora una volta parla di minori. Alla Camera, in occasione dell'adozione della legge che includerà nel nostro ordinamento le norme contenute nello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, il Governo si è assunto la responsabilità,

internazionali: uno dei casi di fronte alla Corte penale internazionale riguarda proprio i bambini-soldato nella Repubblica Democratica del Congo. Speriamo ancora una volta di

più interventi hanno riconosciuto come l'Italia sia un Paese a natalità pressoché zero, anche se negli ultimi anni si è avviato un percorso in positivo in questo senso. Lungi da me voler fare propaganda natalista, ma credo che chi nasce oggi in Italia, molto spesso nasce da genitori non italiani, non cittadini ma soltanto domiciliati, spesso neanche residenti. Occorre tenere presente che la debolezza di tali soggetti è ulteriormente aggravata dalla condizione dei genitori: ripeto, spesso non hanno neanche il permesso di soggiorno, anche se, di fronte alla nostra legge, i minori sono da trattare come gli altri. L'unico piccolo emendamento, o comunque suggerimento, che mi sentirei di fare relativamente all'ordine del giorno G5.200 abbiamo condiviso, in particolare ai punti *g)*, *k)* e *l)*, dove si parla di progetti di ricerca sulla situazione dei minori, dove si parla della possibilità di costituzione di parte civile in procedimenti penali e, nelle modalità di funzionamento presso l'Autorità garante, di una commissione consultiva, è quello di richiedere un'ulteriore particolare attenzione verso la condizione dei minori, dei fanciulli non italiani o comunque provenienti da genitori non italiani, perché possono avere ulteriori difficoltà nel vedere i propri diritti garantiti.

tantissimi bambini in Italia e nel mondo sono e continuano ad essere vittime di violenza: bambini trascurati, maltrattati, usati, abusati. Bambini dall'infanzia negata in mille modi: da una società che propone modelli fuorvianti attraverso programmi televisivi inadeguati, a cui troppo spesso i bambini assistono in solitudine senza guida e controllo alcuno; negata dal fenomeno, ancora nel 2011, dell'abbandono scolastico; negata dall'utilizzo dei bambini da parte della criminalità organizzata; negata dal fenomeno del lavoro minorile; negata dagli abusi sessuali e dalla violenza fino all'assassinio e all'infanticidio; negata dalle guerre e dalla povertà; negata dalle mutilazioni inferte a tante bambine. Purtroppo, l'elenco potrebbe continuare. Il nostro Paese non è mai rimasto a guardare e, attraverso i provvedimenti dei diversi Governi, ha messo in atto tutta una serie di azioni per contrastare ogni tipo di fenomeno, affiancato dal affiancato dal mondo delle associazioni e dal mondo del volontariato. Ma di storie tristi che hanno come protagonisti i bambini se ne sentono ancora tante e lo sappiamo bene. Per un bambino i primi anni di vita sono fondamentali, così come sono fondamentali le esperienze dell'infanzia e dell'adolescenza. Sono questi gli anni più importanti, che plasmano la sua personalità e la persona adulta di domani. I bambini che conoscono la violenza e la sofferenza, durante quelli che per tutti dovrebbero essere gli anni della spensieratezza, conservano purtroppo delle cicatrici indelebili per tutta la vita e molto spesso si trasformano, a loro volta, in adulti vessatori di altri bambini. Come è stato ricordato più volte dai colleghi che mi hanno preceduto, sono trascorsi oltre venti anni da quando è stata approvata a New York la Convenzione sui diritti del fanciullo, con cui gli Stati firmatari - tra cui l'Italia si impegnavano a garantire i diritti del fanciullo attraverso la creazione di specifiche istituzioni incaricate di vigilare sul suo benessere. Oggi anche l'Italia si mette alla pari con gli altri Paesi europei, in cui la figura del garante per l'infanzia esiste da tempo. stiamo discutendo in quest'Aula un disegno di legge che è stato già votato all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento: si tratta sicuramente di un provvedimento di buonsenso, che offre pieno riconoscimento alla figura del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, perché diventi finalmente una

Alla luce della grande assunzione di responsabilità di cui si farà carico chi andrà a ricoprire questa delicatissima funzione, altrettanta responsabilità è richiesta al legislatore nel licenziare la legge, che va a stabilire i requisiti richiesti, i poteri conferiti e le funzioni svolte dal Garante. che l'altro ramo del Parlamento ha approvato all'unanimità il disegno di legge, ma non prima di averlo fatto oggetto, con responsabilità, di un'approfondita analisi, che ha portato all'inserimento di molte modifiche, sicuramente migliorative, rispetto al testo presentato originariamente.

una nota rispetto alla necessità che anche questo ramo del Parlamento possa intervenire con un contributo concreto al perfezionamento del testo, ad esempio per quel riguarda il regolamento di organizzazione dell'ufficio dell'Autorità garante, che sarà adottato di concerto proprio con il Ministro per le pari opportunità.

Solo prevedendo un Garante dell'infanzia che abbia tali caratteristiche si potrà davvero realizzare il dettato costituzionale e le convenzioni internazionali in materia di tutela dell'infanzia. Con lo stesso senso di responsabilità

fondatori, che la Repubblica «protegge (...) l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo», allo stesso tempo esso recepisce quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, che ho citato in precedenza, sottoscritta a New York il 20 novembre del 1989. 1989. Non dimentichiamo poi che la stessa Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, prevede che gli Stati si attivino - ed è quello che sta facendo anche l'Italia - per la promozione e per l'esercizio dei diritti dei minori, attraverso appositi organi. organi. Cari colleghi, quella in discussione oggi in Aula è una legge di buon senso ed è un tassello fondamentale nella difesa dei diritti dei più deboli e dei minori. Certo, non bastano solamente buone leggi per cancellare un fenomeno subculturale; sono indispensabili, ma potrebbero non bastare, quindi non possiamo mai abbassare la guardia in tema di tutela dei minori da ogni forma di violenza, a partire dall'indifferenza che ne è spesso espressione. È necessario - lo sappiamo tutti, ma lo ribadiamo sempre - una cultura amica dei bambini, che li consideri soggetti pieni di diritto e non oggetto di sfruttamento e di mercificazione. Oggi non è più il tempo di battersi con la spada; è tempo di battersi - a mio avviso - a colpi di volontà politica, di precetti di precetti giuridici adeguati. Ed è anche importante che lo spirito, la coscienza e l'esperienza modellino le nostre azioni. Grazie, signora Ministro, per il suo impegno in questa battaglia. Ringrazio anche la collega Serafini, relatrice sul provvedimento, la 1a Commissione e le mie colleghe della Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza. Grazie per la bella pagina politica che oggi stiamo scrivendo e che sarà dedicata a tutti quei bambini che in modi diversi, per cause diverse e in luoghi diversi, si trovano ad avere in comune l'impossibilità di vivere la loro infanzia.

per i loro interventi, ma soprattutto per lo spirito costruttivo con cui hanno affrontato l'esame di questo provvedimento. Il testo, come è stato già detto, è stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati, grazie ad un lungo lavoro che ha visto coinvolte tutte le forze politiche, di maggioranza di opposizione.

alle senatrici del Popolo della Libertà il merito di aver fornito un contributo importante attraverso un ordine del giorno che sollecita la stesura di un regolamento di organizzazione, che renderà sicuramente ancora più efficace

alla relatrice, senatrice Serafini, per il prezioso lavoro di coordinamento e di raccordo svolto per arrivare alla stesura di questo testo. sia una doppia vittoria: da un lato colmiamo un vuoto normativo, rispondendo anche alle sollecitazioni dell'Europa e della comunità internazionale tutta, dall'altro lo facciamo superando le divisioni attraverso un testo che trova d'accordo maggioranza e opposizione. Per questo credo che oggi si scriva una bella pagina per il Paese intero, e in particolare per i diritti dei bambini italiani. *(Applausi)*. «La 1a Commissione permanente, esaminati il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo». parere non ostativo». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno dì legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo. In merito agli emendamenti, esprime parere non ostativo sull'emendamento 3.0.200 e parere di contrarietà semplice sugli emendamenti 2.0.200 e 3.200. Sulle proposte 3.0.201 e 3.0.202, esprime parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla previsione che la partecipazione, a qualunque titolo, del Garante nazionale dei minori, nelle diverse sedi giurisdizionali, debba avvalersi del patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura generale dello Stato. Su tutti i restanti emendamenti l'esame è rinviato».

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione che sull'emendamento 3.0.204, sul quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime poi parere di semplice contrarietà sull'emendamento 3.0.203, nonché sull'emendamento 3.200 (testo 2), limitatamente ai primi tre commi. Ribadisce altresì, in relazione all'emendamento 4.250, la condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già espressa sull'emendamento 3.0.201, relativa all'inserimento di una previsione secondo cui il Garante nazionale dei minori, negli interventi in sede giurisdizionale dovrà obbligatoriamente avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato».

Questo dipende anche dal fatto che tutte le sedi delle pubbliche amministrazioni hanno sede proprio nel centro di Roma. A questo problema se n'è affiancato un altro, che è l'appetito degli immobiliaristi, che ne hanno indubbiamente approfittato: i costi degli affitti di un appartamento romano sono proibitivi per un lavoratore a stipendio fisso con una paga normale. Questo comporta che chi lavora a Roma si deve sobbarcare quotidianamente non pochi chilometri ed il flusso veicolare di chi entra e di chi esce da Roma comporta non pochi disagi per coloro che vi lavorano. Pertanto, pensare a decongestionare il traffico di Roma significa secondo noi soltanto fare il bene di Roma. Venendo al punto, in tantissimi sistemi federati le sedi dei grandi uffici delle grandi amministrazioni dei centri di potere non sono tutte nelle capitali. Se prendiamo ad esempio la Germania, vediamo che Berlino non è sede della Corte costituzionale, la quale ha sede a Karlsruhe,

dello Stato, al punto che, sebbene la Lega ne abbia fatto un tema proprio ed un principio per realizzare un federalismo compiuto, devo ricordare che

che la sede istituzionale dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza non sia ubicata a Roma, ma in una sede che

il precedente *premier* Prodi intendeva organizzare, ma non ha avuto il tempo di farlo, il suo modello istituzionale.

Ciò segnalerebbe il fatto che il Garante nazionale tiene presente sia l'azione comune, sia il fatto che i Garanti regionali sono parte fondamentale dell'azione del Garante nazionale.

questo tema, pur così importante e in grado di eccitare anche certe curiosità e sensibilità particolari, deve essere trasferito in quest'occasione su un argomento che, onestamente parlando, non si presta a questo tipo di accentuazione o di ottica. Noi stiamo varando un istituto che ha una sua peculiarità, una sua importanza e una sua finalità. Sinceramente potrei capire molto di più un dibattito come

cui l'ottimo collega ha inteso motivarlo - voi sapete quanto il modestissimo sottoscritto sia contrario all'ingolfamento in poche megalopoli o in un solo punto di funzioni, strutture, uffici e servizi: per l'amor di Dio, non c'è uno più acceso di me sul decentramento.

Proporrei di sostituire la parola «prevedere» con le altre: «valutare la possibilità di». In questo caso, rimettiamo ad una valutazione successiva

Presidente, mi permetto modestamente di sottolineare al gentilissimo Ministro che comunque non possono andare bene neanche le parole: «a valutare la possibilità perché il testo della legge è molto chiaro. Il testo della legge dice espressamente - lo sottolineo anche a lei, Presidente: "Ferme restando l'autonomia organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorità garante, la sede e i locali destinati all'Ufficio dell'Autorità medesima sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Questo significa che

rispetto a quello che è il testo cogente di un ordine del giorno, è ridicolo. Se vogliamo fare una concessione di questo tipo - non la voglio neanche definire - a un impianto che la Lega voleva in qualche modo introdurre, ciò, tutto poteva avere anche un suo senso, visto l'intervento della senatrice Boldi che faceva prima rilevare come dalle Regioni, in tre Regioni si è già partiti, ci sono possibilità. Però, oggettivamente, o una legge ha un senso, ed è cogente per quello che dice, o non lo ha, e non è cogente. Ma allora, a questo punto, mettiamoci d'accordo. Se vogliamo fare delle regalie (chiamiamole così), facciamole; però, signor Presidente, non possiamo arrivare al ridicolo. Presidente, io eviterei di trascinare su questo provvedimento, che ormai stiamo concludendo, e sul quale abbiamo lavorato per tanto tempo, una polemica, naturalmente con diverse opinioni, come si può ben pensare, sulla questione che è tanto di moda in questi giorni. Io inviterei i colleghi della Lega a riflettere su un punto, che proprio rispetto a questo provvedimento mi pare un po' sbagliato, perché la vera questione dei Garanti

con uffici messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio: e, in questo caso, si può immaginare in quale posto tali uffici possano essere dislocati. Io rafforzerei invece il punto dell'istituzione dei Garanti regionali, che trovo una misura molto importante perché, proprio nell'ottica del federalismo, della capacità e della potenzialità dei territori, questa rete va estesa. Quindi, non è il caso di pensare a un Garante nazionale che abbia sede in altre località, visto che in tali sedi si devono sviluppare i Garanti regionali. Io chiederei, con un po' di buon senso, proprio su questo provvedimento, di evitare una polemica e una posizione che, magari, si potrà assumere su altri punti, ferme restando le opinioni che ognuno di noi può avere.

di quanto richiesto dalla Lega. Colgo ora l'occasione per illustrarlo nei suoi tratti salienti, anche perché il problema posto dal collega della Lega, sulla scia di quanto diceva la senatrice Incostante, è stato, nell'esame della legge, esattamente il contrario, cioè quello di potenziare i Garanti regionali e di sancire la non subordinazione gerarchica dei Garanti regionali rispetto a quello nazionale, il quale, comunque, rimarrebbe in una posizione centrale e, quindi, logisticamente favorevole al raggiungimento della sede da parte di tutti, essendo notoriamente Roma equidistante da tutte le località d'Italia. Detto questo, in realtà, nel nostro ordine del giorno G5.200 sono sono emerse tutte quelle criticità che, da parte dei senatori del PdL ma anche degli altri Gruppi, erano state rilevate, ma che non abbiamo avuto la possibilità di inserire attraverso emendamenti nel disegno di legge che ci era rigidamente arrivato dalla Camera.

all'articolo 3, del Garante nazionale, cercando di dare un ordine e, in particolare, assicurandoci la possibilità che il Garante possa agire in giudizio. Nello specifico, al punto *k)* abbiamo cui il Garante può costituirsi parte civile in procedimenti penali per reati commessi in danno di minori e per intervenire *ad adiuvandum* nei procedimenti civili che, appunto, coinvolgano i minori, con una specifica assolutamente dettagliata. Inoltre, ci è sembrato importante anche sottolineare come debbano essere date forme organizzate di comunicazione, affinché il Garante possa essere adito non necessariamente con il riferimento al numero 114,

esempio, riguardo alle caratteristiche che il Garante deve avere, egli non deve appartenere neanche a sindacati, e non solo a partiti politici. E questo lo abbiamo posto come un requisito che deve essere presente al momento dall'accettazione della carica stessa.

Abbiamo anche tentato di regolamentare le modalità di consultazione, di coordinamento e di collaborazione con i Garanti regionali, ma soprattutto abbiamo anche voluto chiarire il potere di ispezione e di vigilanza del Garante, un punto molto delicato perché si interseca con il lavoro della magistratura, delle pubbliche amministrazioni e della pletora di altri organismi che operano in questo campo. Infatti, il Garante dovrà cooperare con i servizi sociali, le amministrazioni regionali e locali potrà anche fare progetti per la formazione professionale. In particolare, su richiesta della senatrice Baio, abbiamo anche previsto una formazione una formazione omogenea dei curatori speciali dei minori perché, se da un lato il Garante deve tutelare le specificità territoriali dei singoli garanti, deve assicurare un livello minimo di tutela dei diritti omogeneo sull'intero territorio. L'auspicio più importante contenuto all'interno di questo ordine del giorno è che il Garante sia assolutamente autonomo, lontano dalla politica,

Secondo noi dislocare il Garante fuori dalla capitale, che è la massima istituzione, non è proprio fattibile ed è inutile, anche perché, come diceva la collega Serafini, abbiamo istituito

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l'istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza dà attuazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo

evolutiva. L'Autorità che il disegno di legge propone di istituire ha una posizione di indipendenza e un forte rapporto con il territorio, e per essa è prevista anche la consultazione attiva dei bambini e degli adolescenti, oltre che la partecipazione delle organizzazioni riconosciute dall'ONU. Il lungo dibattito che ha preceduto l'approvazione in prima lettura di questo disegno di legge ha comunque consentito l'individuazione di un punto di equilibrio nella costituzione di una figura centrale che tende alla promozione dei diritti di tutti i bambini e degli adolescenti, in sintonia con altre con altre legislazioni europee. Tutti i disegni di legge connessi a questo provvedimento fanno riferimento a convenzioni e a iniziative internazionali in materia di protezione dei minori: dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, alla alla sessione speciale dedicata all'infanzia, svoltasi a New York dall'8 al 10 maggio 2002, dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, all'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli del 1996 e resa esecutiva dalla legge dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, fino all'articolo 10 della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, il cui disegno di legge di ratifica è stato approvato dal Senato, articolo che afferma che le Parti adotteranno le misure necessarie ad assicurare il coordinamento a livello nazionale o locale tra i diversi organismi responsabili della protezione dei bambini,

il testo di questo disegno di legge, che istituisce l'Autorità garante dell'infanzia e su cui siamo chiamati ad esprimere tra poco il nostro voto, è il frutto di un lavoro che non ha evitato il confronto ma che, a differenza delle scene francamente non edificanti viste alla Camera, ha visto prevalere alla fine l'interesse generale sulle piccole dispute tra i Gruppi. La cultura minorile italiana è stata affidata finora a numerose sedi che l'hanno presidiata, dalla giustizia minorile (intesa non solo come magistratura minorile ma anche come servizi del Ministero che le fanno da supporto) ai servizi sociali e alle comunità locali (che si sono attrezzati per garantire ai minori e alle loro famiglie i beni essenziali, i servizi di base); è stata affidata ai servizi specialistici, che hanno preso in carico situazioni delicate di bambini e di ragazzi in difficoltà; è stata affidata ad una elaborazione culturale e professionale delle sedi scientifiche e universitarie, che hanno fatto della cultura minorile italiana un fiore all'occhiello del nostro Paese. Non ci nascondiamo tuttavia che da qualche tempo registriamo, se non una caduta, un allentamento dell'attenzione, poiché assistiamo a troppe situazioni nelle quali persone e gruppi economici senza scrupoli speculano sui bambini in tutti i modi leciti e illeciti, facendoli diventare oggetto o strumento di accumulazione economica o di insano piacere. Assistiamo anche con preoccupazione a fenomeni attraverso i quali i bambini assorbono comportamenti devianti, che vedono rappresentati nei mezzi di informazione. Spesso, infatti, in famiglie che hanno anche difficoltà a curare i bambini, questi vengono lasciati soli ed esposti di fronte alla televisione o ad Internet. Vi è un mondo che aggredisce i bambini, vi è un mondo che va anche oltre il proibito, per arrivare a violare i templi di serenità, di semplicità e di genuinità che sono i bambini. È, quindi, necessario rilanciare la cultura dei diritti dei bambini e degli adolescenti in tutti i suoi aspetti. Questo provvedimento legislativo avrebbe potuto e dovuto rappresentare un modo autorevole per rilanciare questa cultura. Noi abbiamo da sempre puntato in alto, e abbiamo sempre pensato all'Autorità garante, come ad un organismo autorevole, che abbia non solo la capacità di introdurre e di rilanciare l'aspetto culturale, che pure è di straordinaria importanza per il nostro Paese, ma che insieme abbia un qualche potere di intervento e di sanzione. Infatti, Infatti, anche qualora l'Autorità si trovi a constatare che, per esempio, in certi ospedali i bambini ricoverati non possono stare con i loro genitori, o che nel mondo della scuola gli alunni nelle classi sono sovrabbondanti, o, ancora, che vi è una forte dispersione scolastica e non vi è la possibilità di prendersi cura singolarmente di tutti bambini, può esclusivamente segnalare e non intervenire. Come pure quando in televisione o attraverso Internet vengono veicolate situazioni, immagini e modelli che sono distruttivi per il diritto dei bambini a vivere la loro infanzia e l'Autorità garante può al massimo segnalare, ma non sanzionare. Forse avremmo potuto puntare ancora più in alto, sulla scia della positiva trasformazione del Garante in Autorità, decisa alla Camera. Non si trattava solo di una questione nominalistica, ma di una questione di effettività di intervento ed effettività di poteri,

che assorbono tutto dagli adulti, non hanno potere di voto, non hanno potere di rappresentanza politica: semplicemente non hanno potere e non hanno capacità! Ecco perché è necessaria un'Autorità ed ecco perché ci vorrebbe un organismo forte, con reali possibilità di intervento. Tuttavia, è necessario dire in tutta onestà che in questo provvedimento sono state accolte alla Camera numerose altre proposte dell'Italia dei Valori e, tutto sommato, è stato accolto il nostro impianto. Ricordo alcune questioni: la garanzia dell'indipendenza dell'Autorità da tutti i partiti politici; l'attribuzione all'Autorità del potere di vigilanza e di segnalazione, che rende più penetrante la capacità di intervento; la possibilità di chiedere accessi e ispezioni; la Conferenza dei garanti regionali. Già solo il semplice fatto che nel disegno di legge i destinatari della tutela siano indicati come persone di minore età, e non più come minori *tout court*, non è solo una questione lessicale. Il punto è essenziale: da 0 a 18 anni si è persone di età inferiore a quella che dà ingresso alla più ampia e completa gestione dei propri diritti, ma non si hanno diritti minori rispetto a coloro che tale età hanno già compiuto. Questa Autorità è in sintonia con i cosiddetti principi di Parigi e quindi ha quei requisiti di indipendenza e di autonomia che si sostanziano in poteri autonomi di organizzazione, indipendenza amministrativa, assenza di vincoli e di subordinazione gerarchica e sede propria. Tra le sue competenze, c'è quella di promozione del diritto convenzionale europeo e nazionale in tema di diritti delle persone minori di età, di diffusione di buone prassi e protocolli di intesa elaborati dalle Autorità, dagli ordini professionali e dalle amministrazioni. Il testo attuale non contempla modifiche rispetto al testo della Camera: i Gruppi dell'Italia dei Valori e del Partito Democratico (che sempre, insieme alle associazioni, ai magistrati, alle associazioni dei pediatri, hanno lavorato a favore di una politica di promozione e di tutela dell'infanzia) hanno scelto responsabilmente, apprezzando anche l'impegno del ministro Carfagna, di presentare un unico ordine del giorno al fine di favorire la rapida approvazione del provvedimento. E qui permettetemi di ringraziare sentitamente

e ha penalizzato Comuni e Regioni (e dunque non ha certo aiutato i minori, né le loro famiglie), tuttavia consideriamo questo disegno di legge un piccolo rimedio a un *vulnus* pure molto grande. Siamo certi che questa Autorità aiuterà tutti coloro che si battono perché il diritto delle persone minori di età, di qualunque etnia esse siano, prevalga. Noi voteremo a favore di questo disegno di legge perché, grazie al nostro lavoro, pensiamo di consegnare all'Italia, con circa 50 anni di ritardo rispetto al Nord Europa, un provvedimento tutto sommato ben fatto, perché riconosciamo che l'infanzia e le politiche per l'infanzia hanno un valore straordinario e meritano davvero un impegno che sappia andare oltre le ragioni della contingenza politica. Signor Presidente, onorevole Ministri, colleghi, finalmente anche il nostro Paese, a distanza di più di 20 anni dalla Convenzione di New York e di parecchi anni da quella di Strasburgo, rispetta il nostro dettato costituzionale, nonché i precetti contenuti nella Convenzione di New York. Anche noi ci dotiamo di una legge che istituisce questa figura importantissima: un Garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che dovrà lavorare a livello nazionale ed internazionale, poiché oggi i confini dei diritti dei bambini e delle bambine e dei giovani adolescenti non è possibile recintarli dentro l'angusto perimetro nazionale anche per le opportunità che i nostri bambini e i nostri giovani hanno di accedere ad un mercato molto più ampio di relazioni culturali, di relazioni sociali e di relazioni emotive attraverso i nuovi sistemi di comunicazione (vedi Internet e quant'altro) che li mettono nella possibilità oggettiva, anche sfuggendo al dovuto controllo dei genitori e di quanti devono interessarsi di loro, di compiere queste esplorazioni del mondo, che spesso non sono del tutto controllabili e possono anche portare a delle devianze o costituire pericoli oggettivi. Il Garante avrà delle grandi potenzialità di intervento, avrà una grande responsabilità che dovrà condividere con la rete nazionale dei garanti, dovrà lavorare in stretta connessione anche con il Ministro per le pari opportunità oltre che con gli altri Ministeri e la Presidenza del Consiglio, dovrà lavorare soprattutto con le organizzazioni non governative che in questi anni hanno prodotto una mole di lavoro, una mole di dati che sono nella nostra disponibilità, per affrontare un delicato problema, Presidente, che negli anni '70 teneva banco ovunque e dappertutto. I problemi dell'infanzia e dell'adolescenza venivano studiati dai nostri pedagogisti a livello nazionale ed internazionale e la politica se ne faceva carico nei programmi di studio; da troppi anni questo non avviene più. Pertanto, ben venga che il Governo con il Ministro Carfagna si è fatto carico di presentare questo disegno di legge; ben venga che la Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza abbia apportato un proficuo, profondo contributo in particolare tramite la relatrice,

della Presidenza del Consiglio venga fatto di concerto con il Ministero per le pari opportunità. Questa era una lacuna della legge; mi auguro che, inserita semplicemente in un ordine del giorno, non sia presa sottobanco, ma che diventi vincolante. Sta a lei, Ministro, portare avanti questo discorso, perché è nel suo interesse, ma è soprattutto nell'interesse dei nostri giovani e dei nostri bambini. Credo che un lavoro che è durato diversi anni, di cui la senatrice Anna Maria Serafini si era fatta carico in precedenza come Presidente della Commissione, che oggi la Presidente della Commissione attuale ha portato avanti insieme al Ministro, sia un lavoro

che continuiamo a dire minori, perché è giusto (qui ho sentito dire di tutto di più), ma il discorso del diritto soggettivo perfetto del minore è diritto soggettivo perfetto del minore in quanto minore, in quanto va detto che esiste una maggiore età e una minore età. Questo non significa che, essendo minore d'età, il

non ci sarebbe bisogno del Garante. Se c'è bisogno di un Garante, è evidente che è considerata la minore età e non dobbiamo far finta che non esista. Esiste ed è proprio per questo che ha bisogno di accorgimenti legislativi che vadano nel senso del rispetto dei diritti soggettivi perfetti. Signor Ministro, apro una parentesi: spesso nei provvedimenti legislativi «senza ulteriori oneri per le finanze dello Stato». Il diritto soggettivo perfetto che riguarda un minore, giovane o bambino, è perfetto in sé; ma diventa imperfetto quando lo recitiamo dentro il discorso «senza oneri aggiuntivi». Le politiche per l'infanzia hanno dei costi: o ci si fa carico di questo oppure continuiamo a menare il can per l'aia dicendo delle bellissime cose, proponendo anche delle meravigliose leggi, che poi non vengono attuate fino in fondo. Mi auguro che ci sia la consapevolezza, la forza e il coraggio di essere determinanti in quello che qui è stato scritto, perché ce n'è assolutamente bisogno. Un esempio per tutti, Ministro: in questi giorni stiamo assistendo al caso di siti Internet per

pillola di droga, di smerciarla e darla ai loro coetanei. Su questo ci sarà bisogno di intervenire, sì o no? Occorrerà mettere insieme una rete di protezione che, attraverso delle politiche attive del Ministero, del Consiglio dei ministri, del Garante per l'infanzia,

o, se la famiglia non c'è, anche in un ambito sostitutivo della famiglia, con tutte le garanzie che ciò deve comportare, siano effettivamente resi tali. Diversamente, facciamo solo dei bei discorsi, ma poi non arriviamo a conclusioni che possano costituire una risposta ai drammatici problemi che oggi ha ha il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, che è usato, bistrattato, utilizzato dai *mass-media* in tutti i modi possibili e immaginabili, che è usato dalla pubblicità e dalla rete in una maniera così violenta che fa terrore.

carica di essere umano, fatto di carne, ossa e intelligenza, cuore e passione, frutto del suo rapporto genetico con i propri familiari, ma frutto anche di un contesto ambientale che può essere determinante in modo positivo, ma anche in modo aberrante per la sua crescita di futuro cittadino.

dei progetti, delle finalità, degli obiettivi da raggiungere: anche cose semplici, ma una alla volta per favore Signor Presidente, signora Ministro, colleghi senatori, oggi in quest'Aula ci accingiamo ad esprimere un voto importante. Finalmente con questo voto anche nel nostro Paese verrà istituita l'importante figura istituzionale del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, una figura che - è necessario ribadirlo - è presente in quasi tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Per la condivisione unitaria di questa giornata parlamentare voglio ringraziare tutte le senatrici e tutti i senatori, oltre che il Governo,

salvaguardare le specificità dei singoli territori in ragione delle caratteristiche sociali degli stessi. Questo ordine del giorno è stato accolto. Al contrario di quanto si crede, crede, i diritti dei bambini non sono violati esclusivamente in quella parte del mondo che vive in situazioni di grave sottosviluppo, ma anche in quei Paesi che hanno raggiunto livelli di industrializzazione e benessere In tutta la loro gravità si presentano oggi i casi di pedofilia, abuso e violenza sessuale; i genitori evidenziano maggiori difficoltà nell'assolvimento delle competenze delle competenze di cura e di educazione dei figli; le conflittualità intraconiugali e intrafamiliari sfociano in sofferti procedimenti di separazione e di divorzio; sono sempre più evidenti gli episodi di maltrattamento e di violenza intrafamiliare. Per questo rinnovo ancora una volta la gioia di dire che oggi, finalmente, abbiamo una legge che istituisce l'Autorità garante, che tutela i diritti di tutti i minori. Inoltre è importante ricordare come i problemi dell'infanzia, nel mondo industrializzato, segnalano un acuirsi dovuto anche all'ondata dei flussi migratori clandestini. I minori, sradicati dal proprio ambiente naturale, in condizioni di estrema fragilità e povertà, divengono facilmente preda di situazioni di violazione dei diritti fondamentali, dallo sfruttamento del lavoro minorile all'accattonaggio, allo sfruttamento sessuale, all'utilizzo ai fini di microcriminalità. dell'immigrazione e dell'integrazione deve essere affrontato con determinazione, con chiarezza, senza ipocrisia e con grande senso di responsabilità. Infondere un impegno senza tregua nel contrasto di questi fenomeni deve essere una priorità per tutti noi che siamo stati chiamati a rappresentare i cittadini in Parlamento. Pur consapevoli, infatti, da un lato, che le leggi da sole non saranno sufficienti a risolvere questi problemi, dall'altro lato, sosteniamo che proprio grazie all'introduzione di misure di prevenzione programmi mirati e all'impiego di adeguate risorse finanziarie, sarà possibile continuare a sperare di giungere ad una maggiore tutela dei diritti dei minori. I punti cardine sui quali incentrare le politiche di tutela per l'infanzia debbono essere: la conoscenza del problema, il rilancio della scuola come centro di promozione culturale e sociale nel territorio e la centralità del sostegno alla famiglia. La famiglia e la scuola sono certamente i primi ambiti in cui i bambini possono conoscere il valore e il senso della partecipazione. Il Gruppo parlamentare della Lega Nord è convinto che il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, organo monocratico, non soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale, con il potere di verificare l'applicazione e l'osservanza delle leggi nazionali e delle Convenzioni internazionali e di attuare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso la promozione di specifici interventi in materia, rappresenterà uno strumento importante per il contrasto di quelle violazioni dei diritti fondamentali di cui i minori sono vittime. La Lega Nord conduce da anni una battaglia finalizzata alla difesa delle identità culturali e territoriali e dei valori tradizionali e da quando ha assunto la corresponsabilità del Governo del Paese ha sentito, se è possibile, come ancor più irrinunciabile l'esigenza di difendere la famiglia e i diritti dei minori, non a parole ma con atti e scelte politiche chiare. Ci riteniamo anche soddisfatti che il Governo - e qui ringraziamo in modo particolare il ministro Carfagna - abbia deciso di valutare la possibilità di prevedere che la sede istituzionale del Garante nazionale per l'infanzia

*(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo del Partito Democratico esprime piena soddisfazione per l'approvazione di questo provvedimento

un dibattito colto, devo dirlo, anche se è strano per un provvedimento che, probabilmente, quest'Aula non è riuscita ad apprezzare fino in fondo, visto il numero dei partecipanti, per quello che significa. Vorrei riprendere soltanto una questione, che mi sembra la più importante fra tutte. L'approvazione di questo provvedimento non è soltanto l'adempimento di un obbligo internazionale e non è soltanto il compimento di un sistema istituzionale che già vede la presenza del garante per l'infanzia in tante Regioni e amministrazioni locali, ma è qualcosa di più. Lo ha detto la senatrice Serafini, e anche altri

al *mancipium*, che si estendeva a tutti i nati nella famiglia e anche agli schiavi. In questa concezione, che è ancora presente almeno nella sua forma linguistica nel nostro codice civile, si allude ad una minorità dei soggetti che non hanno compiuto i 18 anni che è stata, nel corso delle diverse legislature, dell'avanzare della stagione dei diritti che ha investito profondamente il nostro ordinamento, a poco a poco erosa. Oggi ragioniamo di minorenni e non più di minori. È cambiata anche la denominazione del tribunale specializzato, diventato «tribunale per i minorenni» e non più «tribunale per i minori», come era in origine, perché è andata affermandosi un'idea che oggi accompagna l'attuazione del principio di uguaglianza in moltissimi luoghi del nostro ordinamento e con riguardo a soggetti diversi, che è quella appunto che si misura sull'individuo. Oggi ragioniamo di individuo minore e non più di di soggetti che appartengono alla famiglia. Per questo è stata molto opportuna la citazione fatta dalla senatrice Serafini nella sua relazione nel momento in cui ha letto i versi di Gibran, perché è esattamente così:

del lavoro che ancora ci aspetta, che probabilmente può sembrare altro rispetto a quello che è stato compiuto in questi mesi su questo testo, ma che invece deve partire dallo stesso punto di arrivo. Mi riferisco alle politiche giovanili, che troppe volte, troppo spesso, nella nostra famiglia, nella nostra cultura e nel dibattito politico sono ancora misurate rispetto ai giovani figli. Noi, invece, dobbiamo misurarci con soggetti con individualità piena e la loro uguaglianza dobbiamo assisterla con misure che la traducano nelle pari opportunità di accesso alle risorse economiche, culturali, di diritti sociali. Ora, in tal senso questo punto rappresenta un traguardo prezioso del nostro ordinamento e dovremmo cercare di non dimenticarlo, di non lasciarlo trascorrere, come se esso potesse essere confinato soltanto soltanto a questa occasione importantissima, facendone invece un'acquisizione piena del modo con cui trattiamo tali questioni. Peraltro non è un tema nuovo. Il dibattito politico l'ha conosciuto tante volte e ancora oggi lo riconosce tutte le volte in cui, per esempio, si misura con le politiche fiscali, che fanno fatica a organizzarsi intorno ai soggetti e ad essere misurate in ragione della capacità di promozione che hanno di quei soggetti. Mi riferisco alle politiche fiscali per la famiglia, che noi riteniamo essenziali e fondamentali, ma che non devono mai trascurare il fatto che possono trapassare il dato della promozione delle individualità, dell'autonomia delle individualità e della libertà degli individui.

Onorevoli colleghi, ringraziando il Gruppo per l'onore concessomi nel dichiarare a nome del PDL il voto favorevole sul disegno di legge che, con 1'odierna approvazione, istituisce il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, non voglio esimermi da alcune considerazioni di ordine metodologico. A nessuno sarà sfuggito come, in questa Aula, si sia ritenuto, da parte mia e di autorevoli colleghi del PDL e non solo, di dare un contributo al miglioramento del testo che la Camera ha inviato al Senato, coscienti del lungo lavoro svolto, dal 2009 ad oggi, dall'altro ramo del Parlamento, alla ricerca di equilibri e mediazioni, stante la originaria divergenza tra i punti di vista di maggioranza ed opposizione, ma altrettanto consapevoli che la discussione strozzata presso la Commissione affari costituzionali del Senato, in periodo preelettorale e con un unico relatore di opposizione, non avrebbe reso giustizia a tutti quegli apporti di colleghi della maggioranza che da anni lavorano al tema con competenza, relazionandosi alle realtà sociali che in questo campo operano, proponendo soluzioni normative, le più varie, che certamente non meritavano di essere accantonate *a priori*, fornendo prudenti valutazioni tecniche su un tema che ci appassiona e ci inchioda a responsabilità che devono essere da tutti condivise. Accettiamo quindi, per senso di responsabilità, a questo punto della legislatura, 1'idea che i nostri contributi migliorativi vengano fatti propri dal Governo, che si impegna a recepirli nel regolamento per il funzionamento dell'Autorità garante, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche se alcuni dei temi posti sarebbero stati più propriamente definiti in sede normativa e non in sede regolamentare. Diamo quindi atto a lei, ministro Carfagna, di aver voluto in ogni modo conseguire il risultato positivo dell'istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza che questo Governo, con il contributo di tutti, può oggi iscriversi come tanti altri positivi provvedimenti a favore e a tutela dei soggetti più deboli e meritevoli dell'attenzione della società. Realizziamo oggi un sogno che comincia nei 1989 - come è stato tante volte in discussione ricordato - fatto di disegni di legge, discussioni, audizioni, mozioni parlamentari, emendamenti, *stop and go* ai quali oggi poniamo la parola fine, determinando nel contempo l'inizio di una nuova storia. La figura che si delinea è quella di una istituzione con poteri ampi che - ci auguriamo - non confligga mai con le tante realtà che ruotano attorno al mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, ed anzi ne costituisca il naturale completamento e, dove necessario, coordinamento. motivo per il quale i colleghi senatori di più lunga ed ampia esperienza sul tema consigliavano un *work in progress*. Facile è dare competenze e poteri, molto più difficile è togliere o dirimere i conflitti. Non sarà così - vogliamo crederlo - visti i soggetti cui è rivolta la tutela, ma certo è che colui o colei che andrà a ricoprire questo ruolo avrà puntati i riflettori di tutta la comunità italiana che, pure in sede regionale, si è già organizzata con la istituzione e la nomina dei garanti regionali. regionali. Con estrema onestà credo che, alla luce della istituzione di questa nuova figura, una valutazione vada fatta sul rinnovando ruolo della Commissione bicamerale per 1'infanzia e che in un prossimo futuro si debba ipotizzare una Commissione per l'infanzia in ciascun ramo del Parlamento - così come già avvenuto nel corso della XIV legislatura - che abbia potere legislativo, oltre a quello di indagine, promozione e controllo proprio della Bicamerale attualmente in essere. Credo che il merito di questa legge che ci apprestiamo a votare sia quello di aver delineato, nell'indipendenza e nell'inoppugnabile professionalità ed esperienza, il profilo del Garante italiano per l'infanzia: la indiscussa autorevolezza che dovrà caratterizzare la figura di un Garante che avrà il compito di relazionarsi non solo alle istituzioni dello Stato italiano, ma anche a quelle internazionali. Quale organo monocratico (e nominato) dovrà essere un soggetto capace della massima indipendenza ed equilibrio. Dovrà anche essere una figura capace della più grande sensibilità che si richiede a chi avrà poteri di vigilanza, in alcuni casi di verifica e controllo; che potrà intervenire in giudizio a favore dei minori; che dovrà collaborare, senza invaderne la competenza, con i garanti regionali che non sono ad esso gerarchicamente sottoposti; che dovrà affrontare il tema dei livelli minimi di tutela dei diritti del fanciullo e dell'adolescente (in tema di salute ed educazione, per esempio), propri di un territorio non omogeneo come quello italiano, monitorando e ricercando soluzioni a problematiche che vanno dalla dispersione scolastica, all'abbandono, sottrazione e maltrattamento di minori, disgregazione familiare, all'interferenza dei media nella formazione e nell'educazione del fanciullo, a piaghe emergenti quali bullismo, alcoolismo e droga, *baby*-accattonaggio, lavoro minorile, integrazione di minori stranieri, pedopornografia e prostituzione minorile. Il Garante avrà insomma un ruolo di difesa del fanciullo e dell'adolescente nella società in tutti quei casi in cui la difesa delle tradizionali agenzie appare flebile, debole, non sufficiente, anche se parliamo di genitori. Tutto ciò in un ordinamento giuridico, quale quello italiano, in cui i diritti, e aggiungo gli interessi, dei minori sono al centro della tutela accordata dal diritto penale e civile, in una società in cui la vita, i tempi, gli spazi purtroppo non sono affatto a misura di bambino. a differenza di quanto mi ispirerebbe la mia personale sensibilità, non voglio dar fondo a citazioni, retorica, aneddoti ma mantenere questa dichiarazione di voto nei termini della lucidità e della essenzialità che è richiesta in queste importanti, delicate circostanze. Questo provvedimento, è di tutta evidenza, non nasce infatti sulla spinta dell'emotività ma è frutto di un ragionamento al quale io intendo anche in queste ultime battute dar seguito. Il Garante dovrà avere un ufficio che funzioni; dovrà avere le risorse; dovrà guardarsi dalla politica e dai suoi tentacoli. Dovrà anche ed in primo luogo denunciare tutte quelle incrostazioni alla fine dannose, di progetti naufragati, di risorse malgestite, o di palese incompetenza ed autoreferenzialità che la più bonaria indulgenza ha contribuito a determinare perché a chi agita la bandiera di difensore o amico dei bambini tutto è concesso. Non è così: i bambini, e in questo momento storico più che mai gli adolescenti, hanno bisogno di qualità e di interventi mirati e qualificati. Nutro profonda fiducia sulla futura indicazione che, come la legge prevede, i Presidenti delle Camere vorranno dare al Presidente della Repubblica per la nomina del Garante sintetizzando nella qualità il punto di mediazione. Dichiaro quindi il voto favorevole del Popolo della Libertà a questa legge ringraziando il ministro Carfagna e la relatrice, senatrice Serafini, per la mediazione svolta, e tutti i senatori che trasversalmente hanno dato il proprio contributo, ribadendo l'intendimento della maggioranza di questa Camera a verificare che gli impegni presi dal Governo siano rispettati e declinati, convinta che, ancora una volta, seppure negli angusti spazi di quanto abbiamo potuto fare, il bicameralismo perfetto tanto vituperato, abbia prodotto i suoi migliori effetti.

responsabile, nel solco di una scelta, quella di non intervenire sulla possibilità di miglioramento del testo pervenuto dalla Camera, che rientrerebbe nella logica del sistema bicamerale perfetto, che postula appunto un'esigenza di rivisitazione dei testi nella logica di una reciproca cooperazione. Questo ha fatto il Senato, che oggi compie un gesto di grande responsabilità: privilegia

Con questo vorremmo dare un segnale al Paese, e vorremmo dare un segnale anche al Governo, nell'auspicio che in futuro possano arrivarci dei testi, futuro possano arrivarci dei testi, dopo che l'altro ramo del Parlamento si è pronunciato e ha esaurito ampi dibattiti, che ci diano la possibilità,

Sarei felice se questa convergenza si potesse trovare anche su altri temi: occorrerebbe più buona volontà da parte di tutti, cosa che io mi auguro fermamente. Mi auguro, in sostanza, che l'approvazione unanime di questo testo di legge possa svelenire questo clima, dopo le notizie apprese un'ora fa dalle agenzie secondo le quali degli *hacker* hanno addirittura oscurato dei siti istituzionali. Non è un bel gesto; sono fatto esecrabili, perché l'attacco alle istituzioni è un attacco alla democrazia,

come recita un documento della DIA - come un personaggio poco raccomandabile e facente parte della criminalità organizzata. Dopo la mia denuncia, che risale al 30 aprile - parliamo dunque di quasi due mesi non ho ottenuto nessun tipo di risposta, ma ho avuto continue minacce. In quella casa, dove io non abito, la portiera del palazzo ha già trovato

Francisco. Mi rivolgo a lei, logicamente, in assenza della senatrice Allegrini. In Germania e in Gran Bretagna, per fortuna, da tempo hanno attuato la cosiddetta "capitale reticolare", con il decentramento di varie istituzioni in tutto il territorio nazionale. Ecco, la nostra speranza - lo dico a nome di tutti i colleghi della Lega - è che prima o poi arrivi anche qui da noi questo momento di modernità. **Per

anche per evitare, a proposito di capitali reticolari, che ci troviamo con capitali tentacolari, che alla fine sono peggio di quelle reticolari. Anche di questo bisognerebbe occuparsi, non solo al Sud ma anche al Nord. Detto questo, leggo da un'agenzia che una delegazione di parlamentari del Popolo della libertà ha incontrato il presidente del Consiglio Berlusconi, il ministro dell'ambiente Stefania Prestigiacomo e i Presidenti dei Gruppi

intervenuto chiarendo non tanto che non si possono trasferire i rifiuti ma che per farlo ci deve essere una preventiva intesa tra le Regioni. Ma il tempo in questi casi diventa determinante e fondamentale, per cui si è determinata una emergenza ancora più emergenziale rispetto a quelle che abbiamo già conosciuto. Però, la notizia è appunto di questo incontro, di questa riunione ed occasione. Il Governo, come si legge dal comunicato che i partecipanti all'incontro diramato, si è oggi impegnato a promuovere un intervento istituzionale per consentire la ripresa dei trasferimenti e l'attivazione degli impianti che permettano la più sollecita rimozione dei rifiuti e, finalmente, l'attuazione del nuovo piano regionale sullo smaltimento degli stessi. Ora, il fatto che il Governo promuova degli interventi è un fatto che non coincide esattamente con l'operatività immediata che si dovrebbe determinare. Signor Presidente, qui parliamo di una questione di straordinaria rilevanza.